nel discorso di oggi intendo affrontare gli argomenti di cui si occuperà il Consiglio europeo di questa settimana: pandemia; prezzo dell'energia; gestione condivisa delle crisi; difesa comune; migrazioni e rapporti con Paesi esteri (in particolare Bielorussia e Ucraina). Parlerò anche dei temi in discussione all'Eurosummit: la ripresa economica, l'unione bancaria, l'unione dei mercati dei capitali. L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron, dalle prime indagini molto più contagiosa di quelle finora prevalenti, ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia. I contagi sono in aumento in tutta Europa: nell'ultima settimana, all'interno dell'Unione europea si sono registrati in media cinquantasette casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia l'incidenza è più bassa (quasi la metà), ma comunque è in crescita. Il Governo ha deciso di rinnovare lo stato di emergenza fino al 31 marzo per avere tutti gli strumenti necessari a fronteggiare la situazione. Invito i cittadini a mantenere la massima cautela e a continuare a rispettare le regole che ci siamo dati. I dati di oggi descrivono però un quadro molto diverso rispetto all'anno scorso: il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia è 297.000; mesi fa erano 675.000, nonostante un livello di restrizioni molto maggiore. Le persone ricoverate sono 8.026; il 14 dicembre del 2020 erano 30.860. Negli ultimi sette giorni ci sono stati in media 95 decessi al giorno; nello stesso periodo di un anno fa erano stati 629. Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri. Questo miglioramento è dovuto soprattutto alla campagna di vaccinazione: nell'arco di un anno in Italia abbiamo vaccinato con due dosi quasi 46 milioni di persone e oltre 300 milioni in tutta l'Unione europea. È una mobilitazione imponente, per cui voglio ringraziare il Servizio sanitario nazionale, la struttura del commissario per l'emergenza, la Protezione civile e davvero tutti i cittadini. *(Applausi).*

e oltre il 23 per cento ha fatto anche la terza. Voglio incoraggiare, ancora una volta, chi non si è vaccinato a farlo al più presto e chi ha fatto le prime due dosi a fare la terza appena possibile. Come dimostra un recente studio dell'Istituto superiore di sanità, i non vaccinati hanno un rischio di morire 11 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la seconda dose e quasi 17 volte maggiore rispetto a chi ha fatto la terza dose. Vaccinarsi è essenziale per proteggere noi stessi, i nostri cari, la nostra comunità, ed è essenziale per continuare a tenere aperta l'economia, le scuole, i luoghi della socialità, come siamo riusciti a fare fino ad ora. L'insorgenza della variante Omicron dimostra, ancora una volta, l'importanza di frenare il contagio nel mondo per limitare il rischio di pericolose mutazioni. Non saremo davvero protetti finché i vaccini non avranno raggiunto tutti. I Governi dei Paesi più ricchi e le case farmaceutiche hanno preso impegni significativi per la distribuzione di vaccini gratis o a basso costo agli Stati più poveri. Dobbiamo dare seguito a queste promesse con maggiore determinazione. L'Unione europea ha dichiarato di voler donare 357 milioni di dosi e ne ha già consegnate 134, principalmente attraverso il meccanismo Covax.

Dobbiamo accelerare le consegne e dobbiamo aiutare i Paesi beneficiari a superare i problemi logistici e a migliorare la capacità di somministrazione; questa è l'esigenza più pressante. L'aumento del costo dell'energia è legato soprattutto a cause congiunturali, come la ripresa economica globale e le strozzature negli approvvigionamenti. Questi fattori transitori dovrebbero essere almeno in parte superati nel corso del 2022, con la normalizzazione dei consumi e il superamento dei colli di bottiglia. Tuttavia, i rincari riflettono anche un problema strutturale della transizione energetica. L'espansione delle rinnovabili è ancora incompleta, anche a causa delle esitazioni dei Governi di molti Paesi. Al tempo stesso, per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni a livello globale utilizziamo meno fonti fossili, come il carbone. Il risultato è una dipendenza dai combustibili di transizione, come il gas, con rischi di aumento dei prezzi. Il Governo si è impegnato a definire una chiara traiettoria di decarbonizzazione, con tempi rapidi ma realistici e con obiettivi misurabili. Siamo impegnati a definire un percorso di riduzione delle emissioni a livello europeo che tenga conto della capacità di riconversione del nostro tessuto produttivo. Per aumentare rapidamente la produzione da fonti rinnovabili abbiamo stanziato fondi ingenti e semplificato le procedure amministrative. Nell'immediato la nostra priorità è limitare la volatilità dei prezzi dell'energia che rischia di avere un impatto significativo sui bilanci delle famiglie e delle imprese. In particolare vogliamo proteggere le fasce più deboli della popolazione, che risentono maggiormente di questi aumenti. Da giugno ad oggi il Governo ha stanziato più di 4 miliardi di euro per contenere l'incremento delle tariffe; 1,2 miliardi a giugno, più di 3 miliardi a settembre. Per l'anno prossimo abbiamo previsto di spendere altri 3,8 miliardi e siamo pronti ad aggiungere altre risorse se l'andamento dei prezzi non dovesse stabilizzarsi. Per il primo trimestre del prossimo anno annulliamo gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche domestiche, per le piccole attività commerciali, per le microimprese.

Sempre nel primo trimestre, per i cittadini più poveri e per quelli in gravi condizioni di salute, stanziamo quasi un miliardo per rafforzare le agevolazioni sulle bollette telefoniche. L'Italia è impegnata a trovare L'Italia è impegnata a trovare una soluzione strutturale al problema dei prezzi dell'energia a livello europeo. Penso, per esempio, alla proposta di creare stoccaggi integrati di scorte strategiche di gas; un'iniziativa in tal senso migliorerebbe le capacità di tutti i Paesi europei di far fronte a rialzi dei prezzi improvvisi come quello attuale. Al momento manca un accordo su come procedere, ma è opportuno che il Consiglio continui a occuparsene anche nelle prossime riunioni. Auspichiamo che il terzo pacchetto gas, presentato martedì 14 dicembre dalla Commissione europea, venga attuato rapidamente. Il pacchetto comprende l'acquisto congiunto volontario di stoccaggi strategici da parte degli operatori di trasmissione energetica, una misura che sarebbe utile per far fronte a eventuali rincari futuri. Questa settimana si terrà l'Eurosummit in cui ci confronteremo sullo stato della ripresa economica. La Commissione europea prevede che l'Italia crescerà del 6,2 per cento quest'anno, un tasso superiore a quello dell'Unione europea, pari al 5 Permangono però elementi di incertezza, come la diffusione della variante Omicron e le pressioni inflazionistiche legate anche all'aumento dei prezzi dell'energia. A fronte di questi rischi è giusto confermare una politica di bilancio espansiva per il 2022 che consolidi il sentiero di crescita e punti soprattutto sugli investimenti. All'Eurosummit discuteremo anche del completamento dell'unione bancaria, necessario per rafforzare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria. L'Italia lavora per affiancare ai due pilastri esistenti, il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico, un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Il Presidente dell'Eurogruppo fornirà dei dettagli sullo stato del negoziato in corso a cui l'Italia partecipa e ha sempre partecipato con spirito costruttivo. Nell'Eurosummit discuteremo infine della costruzione dell'unione dei mercati di capitali, un progetto rilanciato grazie al nuovo piano di azione della Commissione europea, presentato nel settembre del 2020. L'azione della Commissione si sta concretizzando attraverso iniziative come la revisione della direttiva Solvency 2 sul comparto assicurativo e il regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine. L'obiettivo è integrare i mercati nazionali dei capitali in un vero mercato unico per aumentare le opportunità di investimento per i cittadini e di finanziamento per le imprese. Al Consiglio affari generali dei Ministri degli affari europei del 23 novembre sono state adottate le conclusioni per mettere a sistema - sono queste le parole Il Consiglio europeo di dicembre inviterà il Consiglio affari generali a proseguire con questo lavoro. Per essere più preparati a eventuali crisi future, vogliamo migliorare le nostre capacità di risposta e tutelare al meglio il funzionamento del mercato unico. Nella prima fase dell'emergenza molti Stati membri hanno cercato soluzioni individuali a un problema comune, lo ricorderete. Penso, ad esempio, alla corsa all'approvvigionamento di dispositivi di protezione, agli episodi di protezionismo sanitario. Nei mesi successivi, però, abbiamo dimostrato di saper collaborare, ad esempio attraverso la centralizzazione degli acquisti dei vaccini. Anche nella risposta alla crisi economica, il coordinamento europeo è stato fondamentale, ad esempio con la creazione del programma Next generation EU. La settimana prossima ci sarà una cabina di regia per approvare la relazione sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel documento sarà illustrato lo stato di realizzazione del Piano, le riforme intraprese, gli investimenti avviati, gli organi preposti al controllo e alla valutazione delle misure. Il Governo farà anche il punto sui 51 obiettivi da realizzare entro la fine dell'anno, che siamo certi di raggiungere entro i tempi previsti. Nel Consiglio europeo daremo, inoltre, un parere iniziale sulla bozza della bussola strategica presentata a novembre dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la La bussola può avvicinarci a un'autentica difesa europea e favorire la costruzione di una cultura strategica comune. Vogliamo migliorare le capacità di gestione di crisi legate a minacce ibride, cibernetiche e alla disinformazione, proteggere al meglio gli spazi geostrategici, oggetto di contestazioni, dai mari allo spazio e migliorare le capacità di risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici, dei disastri naturali, delle emergenze. Inoltre, servirà pianificare meglio gli investimenti per sviluppare le nostre capacità di difesa, incluse le tecnologie emergenti e farlo in modo coordinato, tramite la cooperazione e il supporto tra *partner.* Il negoziato continuerà anche dopo il Consiglio europeo. Intendiamo adottare la bussola strategica a marzo 2022; questa dovrà servire da stimolo per rafforzare la politica estera europea. Servono innanzitutto meccanismi decisionali efficaci in materia di politica estera, di sicurezza, di difesa, a partire dal superamento del principio dell'unanimità che troppo spesso rallenta l'azione europea. Lo stesso vale per i meccanismi decisionali di impiego militare. La capacità europea di pronto schieramento di circa 5.000 unità proposta nella bozza della bussola richiede una struttura chiara e compiti ben definiti. È un primo passo, ma un primo passo importante a cui dovrà seguire, in futuro, una mobilitazione ben maggiore e accompagnata da adeguate risorse finanziarie. Anche i processi di analisi delle minacce e di *intelligence,* da parte delle Agenzie degli Stati membri, devono seguire processi più strutturati e più rigorosi. Dobbiamo tener conto anche delle sfide nell'ambito della sicurezza, che provengono dal Mediterraneo allargato. Bisogna inoltre garantire l'interoperabilità degli strumenti militari europei con la NATO. Un'Unione europea più forte, meglio coordinata e più autonoma dal punto di vista della politica estera è un vantaggio per l'Alleanza atlantica e per il mondo intero. Il Consiglio europeo manderà un segnale di impegno, per rafforzare il partenariato strategico con la NATO: è fondamentale per la nostra sicurezza, anche di fronte a nuove minacce, come quelle cibernetiche. La terza dichiarazione congiunta sulla cooperazione tra l'Unione europea e la NATO, che chiediamo sia negoziata e sottoscritta in tempi rapidi, deve tener conto di queste sfide. Nel Consiglio europeo di domani si parlerà anche di migrazioni. L'Italia pone di nuovo questo tema con assoluta determinazione, anche a seguito del numero elevato di arrivi che ci sono stati in questi mesi. Da luglio gli sbarchi mensili non sono mai scesi sotto la quota di 6.900 e hanno raggiunto un picco di oltre 10.000 ad agosto. Il 14 dicembre le persone sbarcate in Italia quest'anno erano 63.062, nel 2019 sono state 11.097 e nel 2020 sono state 32.919 Al tempo stesso, con l'introduzione delle restrizioni pandemiche, le già sporadiche redistribuzioni tra Paesi europei dei migranti sbarcati in Italia si sono interrotte. L'Italia continuerà a chiedere una gestione condivisa, solidale, umana, sicura. L'Unione europea deve dimostrarsi all'altezza dei propri valori, come l'ha esortata a fare Papa Francesco di recente. Per difendere le vite e i diritti di chi parte per scappare è essenziale promuovere i corridoi umanitari dai Paesi terzi, verso gli Stati membri dell'Unione europea. Non è sufficiente che sia solo l'Italia ad attuarli: serve un chiaro impegno europeo. Dobbiamo rafforzare i canali legali di immigrazione, perché rappresentano una risorsa, non una minaccia per la nostra società. Allo stesso tempo serve una gestione condivisa, rapida ed efficace dei rimpatri. La Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna devono fornire fondi adeguati per la rotta del Mediterraneo centrale e l'Unione europea deve fare di più per negoziare e attuare accordi europei di riammissione e intensificare i rimpatri volontari assistiti. Sul fronte della politica estera, ci aspettiamo che il Consiglio europeo si esprima in modo inequivocabile contro la strumentalizzazione dei migranti da parte del regime bielorusso. L'uso intenzionale dei migranti per scopi politici è inaccettabile. Come ho detto al Primo Ministro polacco durante la sua recente visita a Roma, la risposta europea non è mancata, è stata mirata e concreta. Abbiamo imposto nuove restrizioni nei confronti delle autorità di Minsk e approvato nuove misure di sostegno ai Paesi di arrivo dei migranti: Lituania, Lettonia e Polonia. Occorre anche che questi migranti siano trattati in maniera umana, nel loro passaggio. In queste settimane abbiamo assistito al crescere delle tensioni tra la Russia e l'Ucraina. Il Consiglio europeo deve chiedere urgentemente alla Russia di adoperarsi per ridurle. Dobbiamo rinnovare in modo unanime il nostro sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, come ho avuto modo di esprimere al presidente ucraino Zelensky nella conversazione di ieri. Nelle ultime settimane ci sono state consultazioni da parte del presidente degli Stati Uniti Biden, nel quadro NATO, con l'Italia e con altri Paesi europei, per formulare una risposta. Questa risposta deve partire dalla considerazione condivisa che la diplomazia resta l'unica via per risolvere il conflitto nel Donbass. *(Applausi.

Una soluzione pacifica non può prescindere dall'attuazione degli accordi di Minsk del 2015. Infine, il Consiglio europeo sarà l'occasione per confrontarsi in vista del vertice con l'Unione africana a febbraio. Dobbiamo rafforzare i rapporti con i Paesi africani in ambito multilaterale e con partenariati responsabili e paritari. Tra i temi prioritari ci sono gli investimenti per affrontare la transizione ecologica e la campagna di vaccinazione anti-Covid, che in Africa procede con molte difficoltà. Il Governo auspica che la Commissione e gli Stati membri approvino un pacchetto di misure per l'Africa, anche per accedere alla produzione *in loco* dei vaccini. Nel concludere, voglio ringraziarvi per il vostro contributo e il vostro sostegno. Questi confronti rafforzano l'azione del Governo in Europa e la legittimano ulteriormente di fronte ai nostri cittadini.

Signora Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli colleghi, il suo intervento, signor Presidente, ci consente di entrare in modo molto serio sulle discussioni dei prossimi giorni a Bruxelles, ma questa mattina ella, intervenendo alla Camera, ha voluto - probabilmente come atto molto apprezzato di rispetto verso la tragedia che ha colpito non soltanto il territorio agrigentino, ma tutto il Paese - ricordare i nomi delle vittime. Le siamo grati per questo gesto, per aver consentito al Parlamento di unirsi al ricordo delle vittime,

Nel salutare i suoi ragazzi, andando in pensione, aveva utilizzato parole che giudico straordinariamente toccanti e che mi hanno fatto molto riflettere (come credo a tutte e tutti, in quest'Aula). Egli ebbe modo di dire ai suoi ragazzi: «Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha; non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi; infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non "adattatevi", impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il futuro, siete il presente». Signor Presidente del Consiglio, sarebbe molto bello se il Governo potesse ricordare questo servitore dello Stato, professore del nostro sistema scolastico, con queste parole, che sono uno straordinario insegnamento alle donne e agli uomini giovani, alle nostre concittadine e concittadini più giovani

anche per questo credo che vada chiesto al Ministro della salute di gestire con grande attenzione la comunicazione esterna, perché quello che ha fatto il Governo è il lavoro dei migliori al mondo. In questo 2021 abbiamo vinto vari titoli e sui vaccini siamo stati quantomeno campioni europei, se non in corsa per il campionato del mondo. Sull'economia oggettivamente lei ha ricordato non soltanto la differenza, uno *spread* positivo in questo caso, tra la crescita media europea del 5 per cento e quella del 6,2 che come minimo otterremo.

quindi abbiamo fatto molto meglio di quello che pensavamo di fare. Non lo hanno fatto il Governo da solo o il Parlamento da solo, ma gli imprenditori e le imprenditrici, i lavoratori e le lavoratrici: a tutti loro va il nostro ringraziamento per aver combattuto in modo straordinario in un momento di difficoltà. *(Applausi)*. Tuttavia, il Governo può legittimamente rivendicare questi due risultati. Pertanto, visto che dicembre è tempo di bilanci, diciamola tutta: su vaccini ed economia possiamo girarci indietro e dire che abbiamo fatto un bel lavoro; bravi, complimenti, andiamo avanti. Adesso però la parte positiva è già il nostro passato. Signor Presidente del Consiglio, ho molto apprezzato il suo intervento; per evidenti ragioni di tempo, mi limito a citare alcune delle questioni politiche che nel 2022 questo Governo e questo Parlamento o chi verrà dopo di noi dovranno affrontare. Il primo punto è che non andiamo da nessuna parte, se non mettiamo mano in modo definitivo al patto di stabilità. In quest'Aula nessuno meglio del Presidente del Consiglio conosce la difficoltà del tema, ma c'è il problema che a un certo punto la questione del patto di stabilità ci arriva dritta in faccia. Lei, signor Presidente del con i francesi, nel Trattato del Quirinale, che secondo me è molto importante, un passo in avanti di rilevanza storica, ha sicuramente anche iniziato una discussione preziosa con il presidente Macron lo stesso con il nuovo cancelliere tedesco Scholz. Diciamocela tutta: sul tema del patto di stabilità, il 2022 è l'anno della verità, in una dinamica nella quale avremo qualche difficoltà in più. Non prendiamoci in giro: l'inflazione - basta guardare gli Stati Uniti - è a livelli che non conoscevamo dai tempi di Ronald Reagan. Non importa essere studenti di economia per sapere che era un altro mondo. Abbiamo il problema dell'aumento delle bollette: lo dico perché, in una discussione politica anche tra forze della maggioranza, si è fatto credere che bastasse un piccolo intervento di 248 milioni su una determinata fascia di popolazione per risolvere il problema. La risposta - lo dico anche a una parte dei sindacati che per questo scioperano - è nella notizia che oggi ci ha dato il Presidente del Consiglio - a dire il vero, l'ha data qualche giorno fa

C'è dunque un grande tema e non è che possiamo cullarci sugli allori. La situazione economica ha visto dei passi in avanti straordinari forse bisognerebbe che tutti noi facessimo uno sforzo anche per raccontare che, al di là di quei 248 milioni, negli ultimi cinque anni sull'evasione fiscale siamo passati - cito i dati di ieri del MEF - da 98 a 86 miliardi. Questo per dire che si è fatto un recupero di 12 miliardi, che è una cosa straordinaria, ma contemporaneamente per dire che ce ne sono ancora 86 che sono la vera torta da aggredire. Secondo punto (lo dico con il massimo del rispetto): dal tema della NATO e dell'Unione europea, su cui il Presidente ha speso parole importanti qualche istante fa, istante fa, non si scappa. Ricordo anche in quest'Aula i sorrisini, quando Emmanuel Macron disse che la NATO era in una condizione di morte cerebrale. Aggiungo che per me non è cerebrale, ma morte pura, e possiamo soltanto cercare di rilanciarla. Mi auguro che il Governo e il Parlamento, quali essi saranno, nel 2022 lottino per un segretario generale della NATO perché penso che sia importante portare i valori che il Presidente ha citato oggi nella discussione europea (intendo un italiano che ami Bruxelles, ci siamo capiti). Terzo e ultimo punto che mi sento di sottolineare è il tema dell'immigrazione. Il 2021 è stato l'anno in cui, plasticamente, si è dimostrato - numeri alla mano - che due immigrati di seconda generazione (in un caso, neanche di seconda generazione), in Germania, venendo da un Paese fuori dell'Europa, la Turchia, hanno salvato il mondo col vaccino:

il tema dell'immigrazione finalmente dev'essere affrontato non soltanto come emergenza, ma anche e soprattutto come opportunità: lo ha detto lei, Presidente, e noi siamo con lei. So, Presidente, che questi argomenti richiederebbero molto tempo e approfondimento, ma grazie per quello che sta facendo. giustamente preoccupato per quello che succederà nelle prossime settimane, è naturale e fisiologico. Credo che si possa guardare in positivo e dire che l'appello che ha fatto la *leader* di Fratelli d'Italia a eleggere un patriota al Quirinale sia un'ottima idea. Noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo. Patriota è stato Carlo Azeglio Ciampi, patriota è stato Giorgio Napolitano e patriota è stato Sergio Mattarella, cui vanno il nostro deferente saluto e un grande ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni.

Presidente, signor Presidente del Consiglio, vorrei fare una riflessione complessiva sul rapporto tra l'Italia e l'Europa in questo anno che sta per chiudersi, il 2021. Secondo me, ci sono state tre dimensioni ugualmente importanti e tutte e tre chiaramente nella direzione positiva. Primo: si è rafforzata la posizione dell'Italia in Europa. Secondo: si è rafforzata la posizione dell'Italia nel mondo, grazie alla Presidenza italiana del G20. Terzo: si è rafforzata la posizione dell'Europa in Italia e nella percezione degli italiani. In particolare, i successi dell'Italia sono ovviamente dovuti al prestigio personale e alla riconosciuta autorevolezza del presidente Draghi, alla qualità del Governo e all'attenzione crescente - mi sembra - che il Parlamento e l'opinione pubblica prestano a queste questioni, vissute sempre di più come grandi fattori interni di evoluzione della società, dell'economia e della politica italiana. Si è trattato quindi di grandi meriti del Governo in subordine, del Parlamento - e anche di maturazione dei frutti di opere precedenti, come nel caso del trattato tra l'Italia e la Francia. Trovo molto significativo che questo trattato, che rafforza la coesione tra i nostri due Paesi, venga nel momento in cui non in chiave antagonistica, ma in chiave - io trovo - perfettamente complementare, è uscito il contratto di coalizione del nuovo Governo tedesco, che ha molti valori in comune

si arriva a parlare con maggiore scioltezza e con minore dose di riserva mentale reciproca persino di temi delicatissimi come sovranità e patriottismo. Ormai è chiaro a tutti che esiste anche una Patria europea accanto a quella - per noi - italiana ed esiste solo la via europea in determinati campi, in altri no, per conseguire effettivamente una sovranità efficace per l'Italia e per gli altri Paesi. Auguro vivamente a tutti noi che le grandi sfide che ci sono per il 2022 - il senatore Renzi ne ha elencate alcune molto grandi - possano essere affrontate con tutta la dose di dibattito necessario, ma nello spirito che, secondo me, si sta formando e del quale naturalmente la presenza attiva e vigorosa del presidente Draghi è un importante ingrediente. Concludo dicendo che il prossimo anno sarà importante, delicato e forse un po' più controverso del 2021, perché ci saranno costruzioni in cantieri nuovi

che, come sappiamo, sono stati sospesi, ma hanno mostrato anche la necessità di un aggiornamento abbastanza radicale. Spero che anche dal lato del Parlamento, signor Presidente del Consiglio, si possa collaborare,

Presidente, colleghi, la Commissione europea il 13 ottobre 2021 ha detto che la migliore assicurazione contro l'aumento dei prezzi è la transizione verso l'energia cosiddetta pulita, efficientamento energetico ed energie rinnovabili. L'aumento dei prezzi dell'energia riguarda tutti, anche se ne risentono soprattutto le persone in condizioni di povertà energetica e le famiglie a reddito basso e medio-basso. Nel 2019, infatti, circa 31 milioni di persone non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione ed è quindi chiaro che sono necessarie misure immediate a sostegno delle categorie più vulnerabili, come lei ha ben detto, Purtroppo il gas naturale riveste ancora un ruolo importante nel *mix* energetico dell'Unione europea e anche nel nostro Paese e gli esiti della COP26 non sono incoraggianti quanto all'abbandono delle fonti fossili. Nel 2021 gli effetti della pandemia hanno condizionato gli scenari energetici internazionali, ma la buona notizia è che la domanda di energie Un'altra buona notizia riguarda la minore dipendenza del nostro Paese dalle fonti di approvvigionamento estere, un aumento peraltro, ancora una volta, della produzione di energia rinnovabile, che rappresenta circa il 70 per cento del totale della produzione italiana. Velocizzare il processo di transizione verso le energie rinnovabili significa anche intervenire concretamente e velocemente nell'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Va chiarito ai cittadini che l'esborso da parte dello Stato di soldi pubblici per finanziare ancora l'energia prodotta da fonti fossili significa distruggere l'ambiente, la salute e l'economia, quindi il nostro futuro. Quanto poi allo sviluppo delle energie rinnovabili marine, ricordo il gravissimo ritardo (di ben nove mesi) nella pianificazione dello spazio marittimo e quindi a favore del piano per la riapertura delle trivelle, sia in mare sia a terra, per l'estrazione del gas, che diventa di fatto preminente rispetto allo sviluppo dell'economia circolare del mare, che dev'essere sostenibile e integrata rispetto a tutte le politiche relative al turismo, alla pesca, ai trasporti,

ricchissima). Le chiedo di porre attenzione al *mix* energetico, di cui il Parlamento ancora non ha conoscenza, perché non abbiamo ancora l'aggiornamento del Piano nazionale per l'energia e il clima. clima. Non possiamo fare quindi un atto di fede, ma abbiamo necessità di comprendere e di portare avanti, secondo quello che ci chiede la Costituzione, un'azione di controllo di quello che fa il Governo.

signor Presidente del Consiglio dei ministri, membri del Governo, qualcuno ieri, durante un momento importante della vita parlamentare, parlando e ragionando dell'attuale momento legato all'energia, ha ha dato una definizione che ho apprezzato molto: da qui all'ambizioso obiettivo della neutralità climatica, dobbiamo vivere. Mi sembra che questo sia un bel manifesto sul quale poter ragionare. Si aggiunga a questo la dichiarazione del vice presidente esecutivo per il *green deal* europeo, Timmermans, per cui la responsabilità del caro energia è legata solo per un quinto al processo di decarbonizzazione.

lo scarso valore del *mix* energetico in Italia e, soprattutto, la grandissima dipendenza dalle importazioni, nonostante l'incrementato ricorso alle rinnovabili, che non riesce a colmare il *gap*. La crisi energetica, presidente Draghi, sta colpendo i costi di approvvigionamento di gas naturale ed energia elettrica e ha un orizzonte di difficile previsione. Anzi, a detta di molti analisti, potrebbe esserci un ulteriore *shock* dell'andamento dei prezzi, per fattori esogeni alle normali dinamiche di mercato e attualmente poco prevedibili. Al fine di essere in grado di contenere con prontezza eventuali e improvvisi rialzi del costo della componente energetica, occorre, a mio e a nostro avviso, ampliare la dotazione del margine di manovra dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente almeno a tutto il primo semestre 2022, se non oltre. Signor Presidente, lei faceva riferimento nel suo discorso al fatto che, da giugno ad oggi, il suo Governo ha già stanziato oltre 4 miliardi e si appresta ad aggiungere altre risorse per il raggiungimento dell'obiettivo, non ultimo l'annullamento degli oneri di sistema per le utenze elettriche domestiche e per le piccole attività e le microimprese. Le dico che va molto bene,

Ha poi continuato dicendo che l'Italia è impegnata a trovare una soluzione strutturale al problema dei prezzi dell'energia a livello europeo. Perfetto, ne sono molto contento. La sua autorevolezza in Europa è stata richiamata già più volte, quindi sono molto fiducioso in questo. Le chiedo pertanto di impegnarsi fortemente, affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico. A questo proposito, serve assolutamente rivedere l'esclusione dai progetti di interesse comunitario, in forza del regolamento TEN-E, del raddoppio del TAP, infrastruttura che invece è fondamentale per il rafforzamento della capacità di trasporto del gas in Italia, per la diversificazione degli approvvigionamenti e per ridurre i costi di approvvigionamento del gas. Quando parliamo di raddoppio, ovviamente lo facciamo non dal punto di vista ambientale, come impatto, ma della potenza delle emissioni e della quantità di gas da ricevere. Non ultimo, occorre definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca le regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti del gas. La regolamentazione degli stoccaggi e i relativi profili di utilizzo - e questo lei e il suo Ministro lo sapete perfettamente - immagino sia, per voi come per noi, la condizione essenziale per la nostra sicurezza energetica. Presidente Draghi, mi preme altresì chiederle di sostenere l'aumento della capacità estrattiva dei giacimenti esistenti in Italia, anche perché non si capisce come mai siamo gli unici a non utilizzare la nostra totale possibilità, magari poi acquistando energia elettrica dalla Francia, 15 per cento, derivante esclusivamente dal nucleare, sul quale finalmente si sta aprendo un dibattito. Mi chiedo poi se siamo proprio sicuri che sia una buona idea litigare con la Russia, soprattutto alla luce del fatto che Mosca è il principale fornitore europeo di gas e sta onorando tutti i contratti di approvvigionamento. Signor Presidente, è illogico voler colpire chi sta rispettando gli accordi. Mi permetto Mi permetto inoltre di far presente come la proposta di acquisto comune europeo di metano sia piena di incognite operative e presupponga comunque un ruolo determinante di Mosca. Occorrerebbe piuttosto muoversi subito con decisione per rimuovere il meccanismo del *panking* e tariffario del gas. La realizzazione di un mercato unico europeo è esposta al rischio di comportamenti opportunistici dei singoli Stati membri. Non sarebbe la prima volta che accade e probabilmente non sarebbe neanche l'ultima. La competitività del gas è spesso condizionata dalle decisioni delle autorità estere, che possono agire in maniera discriminatoria per favorire i loro consumatori, a discapito degli altri Paesi.

grandi. Apprezzo la perplessità che il Governo ha posto sullo stop alle auto a combustione al 2035. È evidente che forse non c'è neanche un miglioramento dal punto di vista ecologico, ma di sicuro perderemo 70.000 posti di lavoro. Signor

Presidente, signor presidente Draghi, ammesso le interessi ciò che è interesse degli italiani che non l'hanno votata, ma sono da lei, loro malgrado, rappresentati nel Consiglio europeo, sono a portarle qualche voce che proviene dalla riserva indiana in cui ha confinato parte della società che prudentemente e con ogni santa ragione non ha ritenuto di fare le scelte da lei caldeggiate e raccomandate in merito alle vaccinazioni di massa, in assenza di sufficienti studi clinici a breve, medio e lungo termine. Le chiedo conto intanto della fondatezza giuridica e fattuale della proroga di uno stato d'emergenza oltre i limiti fissati dalla Costituzione. Lo stato d'emergenza porrebbe i suoi presupposti sul contenimento dell'epidemia da Covid-19, Covid-19, che ha un indice di mortalità dello 0,2 per cento, in presenza oltretutto di un 10 per cento dei posti in terapia intensiva occupati. Lo stato d'emergenza si fonda su interventi militari, ma per fare cosa? La guerra a un microbo o a onesti cittadini inermi, colpevoli solo di aver compreso i vostri inganni ed esservisi sottratti? Innanzitutto, prima di parlare nel Consiglio europeo di misure economiche, dato che le Nazioni non sono aziende - nemmeno quella da lei rappresentata lo è pretendiamo che ribadisca il diritto all'inviolabilità delle persone, diritto umano riconosciuto da tutte le convenzioni internazionali sottoscritte anche dall'Italia, oggi misconosciuto proprio nel cuore della civile Europa e qui in Italia, in particolare, grazie alle misure da voi portate avanti. Pretendiamo che lei chieda che vengano rimossi tutti i conflitti di interesse in capo alla Commissione europea e agli organi di autorizzazione dei farmaci. Pretendiamo che ci dia conto degli impegni assunti a livello internazionale per cui ha esteso unico caso anche in Europa - l'obbligo vaccinale sul posto di lavoro, con sanzioni incostituzionali, che privano i sanzionati del sostentamento,

circa 30.000 morti nei 27 Paesi dell'Unione europea in concomitanza con le somministrazioni di questi farmaci e 3 milioni di eventi avversi. Per la Costituzione italiana, ma anche per la Carta di Nizza, per il codice di Norimberga e la Convenzione di Oviedo nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario che può condurlo all'invalidità e alla morte, fosse anche il farmaco più socialmente utile mai realizzato, e lei sa benissimo che questi farmaci non assolvono nemmeno alla funzione di limitare i contagi, poiché anche con le terze dosi ci si contagia. Parliamo quindi solo di grandi affari per le case produttrici, ma forse era a questi impegni che faceva riferimento in premessa al decreto-legge n. 172 del 2021; forse è a questo che si deve la compressione dei diritti contenuti nei primi articoli della Costituzione: a volgari accordi commerciali. A questo si deve la guerra che ha dichiarato al popolo italiano, distruggendone il tessuto sociale e produttivo? Ma lei chi rappresenta veramente qui e nel Consiglio europeo? La proporzione tra la violenza e l'abuso con cui sono imposti questi farmaci e la loro efficacia è sotto gli occhi di tutti, anche dei più ciechi, ottenebrati dalla propaganda pagata con soldi pubblici. Non scambi però la rassegnazione di alcuni con il favore per queste misure liberticide ed esiziali per il popolo italiano. Per quanto ancora, col portafoglio vuoto, gli italiani continueranno a credere alle menzogne dei TG, che annunciano magnifiche sorti e progressive, che nessuno vede all'orizzonte, almeno di noi comuni mortali? Pretendiamo che lei non prenda accordi per nessun progetto sociale ed economico che riguardi il nostro Paese che travalichi i limiti imposti dalla Costituzione italiana, su cui ha giurato. Pretendiamo che ai medici sia tolto lo scudo penale, perché il cittadino sano, trasformato contro la sua libera determinazione in paziente, curato in serie, non può accollarsi pure la responsabilità di un trattamento su cui non sussistono sufficienti informazioni scientifiche per valutarne efficacia e rischi (rischi che le case farmaceutiche non si accollano e di cui uno Stato che impone obblighi non può non farsi carico per intero). Pretendiamo che riferisca in Consiglio europeo che, con un virus che ha una letalità dello 0,2 per

*(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, solo due mesi fa ci trovavamo in quest'Aula ad affrontare il problema del caro energia. Dal dibattito emersero palesemente due elementi: il primo è che l'aumento sarebbe persistito ancora per molti mesi, con conseguenze economiche molto preoccupanti, sia dal lato dell'inflazione, sia per il pericolo di un rallentamento, se non addirittura di un'interruzione, della ripresa; il secondo è che le cause intrinseche, strutturali di questo aumento derivano dalla struttura del sistema energetico europeo, fortemente dipendente dall'importazione del gas. L'Unione europea, pur disponendo di un sistema di infrastrutture di importazione diversificato, non può sottrarsi alle dinamiche globali, non domina le dinamiche degli aumenti di prezzo. In quell'occasione avevo sottolineato quanto questo forte aumento riguardasse tutti gli Stati, anche quelli più nuclearisti, legati comunque alle stesse regole di formazione dei prezzi sui mercati internazionali, tanto da rendere palesemente antieconomica qualsiasi ipotesi di riapertura al nucleare (e sul nucleare tornerò a sprazzi nei prossimi minuti). A distanza di pochi mesi, possiamo affermare che il quadro non è cambiato, anzi, è addirittura peggiorato: le attività produttive e le famiglie sono in forte difficoltà e abbiamo poco tempo. Tra le cose che avevamo condiviso nel dibattito scorso, vi è l'opinione comune e trasversale, indicata anche nella comunicazione 660/2021 della Commissione al «La transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere sull'acceleratore». Per energia pulita ovviamente si intendono le fonti rinnovabili, che sono più veloci, più economiche e più controllabili. esprimiamo apprezzamento rispetto alle posizioni assunte in Europa, nel Consiglio energia, con il "non-paper", in cui abbiamo chiesto che il *market design* elettrico sia adattato al ruolo centrale delle energie da fonti rinnovabili nell'orizzonte 2030.

alla produzione di auto endotermiche entro il 2035, che darà una forte spinta verso l'elettrificazione e un grande stimolo alla conversione del settore produttivo, che la politica deve accompagnare, Importanti sono naturalmente gli interventi adottati dal Governo in questi giorni, che saranno inseriti nella manovra, per calmierare gli aumenti dei prezzi (interventi quindi necessari e utili, ma non risolutivi). Gli aumenti dei costi della bolletta vanno infatti presi di petto prima che il sistema produttivo entri in cortocircuito. Su questo siamo tutti d'accordo; ciò su cui siamo meno d'accordo sono le soluzioni che devono essere individuate per affrontare e calmierare strutturalmente tali aumenti. Al di là quindi delle ipotesi nucleari,

accumuli e la concretizzazione di una vera concorrenza nel mercato dei servizi elettrici, purtroppo incagliati nei ritardi di produzione delle norme. Sono tanti gli operatori da tempo in attesa di provvedimenti normativi che non arrivano.

È di ieri la notizia che conferma lo slittamento e il conseguente ritardo di un anno delle nuove regole su trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso di energia elettrica prelevata, funzionale a consentire la successiva immissione in rete, cioè quella relativa agli accumuli, e i servizi di generazione. del Consiglio, quello che le voglio dire in linguaggio non politico è che non è un problema di tecnologie, ma di norme che non riusciamo a produrre. Qui facciamo tanti bei discorsi ed emaniamo anche buone leggi, ma poi ci sono i classici sassolini che bloccano gli ingranaggi: è su questo che il Governo deve stare più attento.

parliamo infatti di speculazione finanziaria e su questo so che lei è una persona estremamente competente. Sono sicuro che il suo Governo farà tutte le opportune verifiche per intraprendere eventualmente le conseguenti azioni necessarie. Lei ha detto che il Governo è impegnato a definire una chiara traiettoria di decarbonizzazione e un percorso di riduzione delle emissioni a livello europeo che tenga conto della capacità di riconversione del nostro tessuto produttivo, aumentando rapidamente la produzione da fonti rinnovabili. dichiarato che gli stanziamenti per calmierare gli aumenti non possono andare avanti all'infinito, ma occorre trovare soluzioni strutturali e fare una riflessione sul meccanismo del prezzo dell'energia. È ciò che avete già provato a ipotizzare in Europa al fine di cambiare il meccanismo del prezzo dell'energia: questo va fatto. Plaudo anche al tentativo di realizzare finalmente una comunità dell'energia, quindi gli stoccaggi in comune, anche se su base volontaria: questo mi sembra un passo decisamente in avanti e sarebbe ora che l'Unione europea facesse l'Unione europea; su questo ci trova perfettamente allineati. Contro il caro energia quindi non c'è un'unica soluzione, ma una pluralità di soluzioni. Noi abbiamo una cassetta degli attrezzi pronta, dobbiamo accelerare su questo e passare dalla volontà di fare al fare. Se veramente questa è la strada che il suo Governo vuole battere, da parte nostra avrà pieno supporto. Un ultimo doveroso passaggio, signor Presidente, lo faccio sulla tassonomia verde europea. tale riguardo, ribadiamo come MoVimento 5 Stelle quello che abbiamo già espresso più volte - anche formalmente abbiamo depositato una mozione a inizio agosto sottoscritta da tutto il nostro Gruppo parlamentare - ossia - ossia la necessità che il suo Governo intraprenda ogni opportuna iniziativa presso le istituzioni europee per escludere le attività relative all'energia nucleare e al gas *(Applausi)* da quelle che si possono definire sostenibili. Viceversa, vorrebbe dire che incentiviamo strumenti che sono persino dannosi, perché allontanerebbero sia la finanza privata sia il denaro pubblico da investimenti realmente virtuosi e dagli obiettivi climatici che ci siamo posti e che servono naturalmente per far sopravvivere il genere umano, mentre porterebbero ancora denaro su tecnologie che hanno dimostrato di non essere la soluzione.

già sappiamo non essere la scelta più giusta da fare o addirittura a tecnologie che creerebbero ulteriori problemi con cui dovremmo poi confrontarci. Disponiamo di risorse cospicue, destinate alla transizione ecologica dall'Europa; non indirizzarle verso...

per cultura e per carattere non sono una catastrofista; anzi, mi si prende sempre in giro perché sono una persona che tende sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche per trovare la forza di recuperare quello che manca e renderlo veramente pieno. Ho avuto questo atteggiamento anche rispetto all'Europa, ma le devo confessare, presidente

con un'insopportabile retorica, e proprio da quelli che oggi si girano dall'altra parte, accettiamo che anche dentro i confini dell'Unione si parli di di tenere fuori, di respingere. Ebbene, non riesco a capacitarmi: come è possibile che un continente di 500 milioni di abitanti chiuda fuori 6.000, 7.000, 8.000 disperati sul confine Bielorussia-Polonia, e anzi li affoghi con gli idranti, che mandi l'esercito? Parliamo di poveracci che

è mai possibile? È mai possibile? Se potessimo con un drone guardare dall'alto vedremmo un continente con tutti i suoi problemi, ormai pieno di muri: si pensi ai 150 chilometri del muro ungherese, per esempio, o alla barriera di Ceuta e Melilla in Spagna oppure al Passo di Calais o a Ventimiglia. Ecco, credo che, mentre andiamo avanti dal punto di vista economico - della qual cosa sono contenta e la ringrazio molto - stiamo perdendo per strada i valori che continuiamo a sbandierare, ma che nella pratica calpestiamo. Insomma, è come se in Europa, signor Presidente del Consiglio, stia morendo persino la pietà,

Mi si dice che la Libia non è all'ordine del giorno del Consiglio - è vero - ma, sa, presidente Draghi, è all'ordine del giorno della realtà, perché l'accordo fatto sulle elezioni entro Natale di tutta evidenza salterà, non verrà rispettato; non c'è neanche la legge elettorale, quindi ce ne dovremo occupare. Spero, come lei ha detto, che finalmente ci renderemo conto che, con una buona accoglienza, queste persone possono essere un *asset*

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghe e colleghi; signor presidente Draghi, come è cambiata la percezione dell'Europa con lo scoppio della pandemia. Ricordo alcune definizioni tipo la matrigna, il tiranno o addirittura la sanguisuga; oggi invece l'Europa è vista come una comunità solidale che riesce a condividere addirittura il debito pubblico dei singoli Paesi per sostenere le economie e per rispondere ai gravi danni che derivano dalla pandemia.

ha avuto la lungimiranza di inserire alcuni punti che da troppi anni sono sul tavolo europeo, nodi che non vengono sciolti. Lei ha parlato di politica comune di difesa, di politica comune estera e di sicurezza. Mi permetta di aggiungere, presidente Draghi, il riferimento alla politica comune fiscale, che genera disparità e concorrenza sleale tra i Paesi membri, persino con la delocalizzazione di molte imprese. Noi, nonostante questo, presidente Draghi, continuiamo a credere che l'Europa vada rafforzata per poter far fronte alle sfide globali. Mi permetta di esprimere, presidente Draghi, a lei e al suo Gabinetto, un apprezzamento per il fatto che Paesi autorevoli dell'Unione europea hanno preso l'Italia come modello della lotta al Covid. Questo è un plauso che merita l'intero suo Gabinetto e la sua persona. Tutto questo inorgoglisce il senso patriottico che ciascuno di noi ha nella sua cultura e nella sua formazione. In questo periodo si è abusato un po' di questa parola; ha ragione la presidente di Fratelli d'Italia, onorevole Meloni, quando dice che è in corso una polemica stucchevole sulla definizione di patriota. Mettiamola da parte. La domanda però è la seguente: come difendiamo al meglio gli interessi nazionali nello scacchiere non solo europeo, ma anche globale? Questa è una domanda. Mi si permetta anche una provocazione non tanto ingenua, ma priva di pregiudizi; l'Europa a guida sovranista tutela al meglio gli interessi dei singoli Stati membri e, per quanto ci riguarda, gli interessi particolari dell'Italia? Ecco, noi non lo crediamo, noi crediamo che ci voglia più Europa, più unità e più solidarietà tra i Paesi. Signor Presidente del Consiglio, vogliamo anche chiudere questa parentesi prendendo la definizione di patriota mi dispiace ma non convengo con l'intervento della senatrice Bonino. Forse talvolta ci dimentichiamo che i Padri fondatori hanno voluto questa unione non solo come aggregazione di interessi economici, volendola fondare invece su un pilastro di condivisione di valori e di principi. Vi è troppa timidezza, presidente Draghi, lo dica al Consiglio europeo, nel difendere le nostre radici giudaico-cristiane.

ma nella direzione di non garantire l'inclusione culturale e sociale, senza difendere la propria identità e le proprie radici. *(Applausi)*. Vogliamo denunciarlo a chiare lettere, signor Presidente. Presidente. Arrivando ai punti salienti della sua relazione, come non condividere la parte in cui lei dice che bisogna rimuovere su alcuni temi strategici l'unanimità, un ostacolo dirimente rispetto alla competizione globale, che permette di alimentare una narrazione in cui l'Europa è ferma per un vincolo francamente assurdo ed anacronistico. Su alcuni temi strategici si passi alla maggioranza relativa o alla maggioranza qualificata, eliminando l'unanimità. Su alcuni passaggi, Presidente, tutti gli indicatori economici sono positivi. Non dobbiamo però abbassare l'attenzione, perché, come lei stesso ha enunciato, il tema è il rischio di inflazione

speriamo che si attui quello che lei ha detto, ovvero il terzo pacchetto del gas: è evidente che un contraente che rappresenta 500 milioni di cittadini al tavolo delle contrattazioni con i vari servizi di erogazione del gas ha un peso contrattuale superiore se parla con un'unica voce, rispetto a chi magari va da solo a trattare. Presidente, mi permetta di fare, in L'Europa ha una cultura che le permette di affrontare crisi di questo genere attraverso la fermezza, certamente, ma anche attraverso il dialogo. Noi non siamo il gendarme del mondo,

presidente Draghi, complimenti a lei e al suo Governo per come sta conducendo la lotta contro il Covid. Siamo tra i migliori al mondo, siamo i migliori in Europa. una realtà completamente diversa rispetto a quella che ci aveva lasciato il Governo Conte-*bis*, ma noi non avevamo dubbi nel momento in cui, con il nostro *leader* Matteo Salvini, abbiamo deciso, da protagonisti, di dare vita e di sostenere questo Governo. Siamo i migliori perché nella campagna di vaccinazione siamo tra i primi, siamo i migliori anche per quanto riguarda i contagi: ci sono meno contagi in Italia che in tutta Europa, con un'incidenza uguale

le felicitazioni più grandi per il nuovo incarico che ha ricevuto a capo del Comando operativo vertice interforze (COVI), un incarico assolutamente meritato. Mi si consenta anche di dire grazie a tutti gli italiani, un popolo che si è dimostrato ancora una volta meraviglioso.

Dico anche grazie a tutti quegli italiani che non intendono vaccinarsi perché la vedono diversamente, ma dico anche che a un certo punto, in quest'Aula, Presidente, bisogna anche tracciare una linea, bisogna anche dirsi delle cose con franchezza. esempio bisogna dire basta a coloro i quali portano avanti, con minacce e con violenza, una campagna di odio contro i vaccini e contro coloro i quali sono a favore dei vaccini. A queste persone bisogna dire basta, perché non possiamo stargli dietro, perché una cosa è vederla diversamente, con queste persone ci si confronta, si mettono sul tavolo le idee diverse, ma altra cosa è minacciare, altra cosa è esercitare violenza. Anche per questo, nei suoi confronti, presidente Draghi, esprimo tutta la solidarietà per le minacce che ha ricevuto; lo faccio nei confronti del governatore Fedriga, che è impegnato a governare la sua Regione e a fronteggiare, come tutti i governatori, questa maledetta pandemia e si vede costretto a girare scortato. Siamo alle porte del Natale.

perché è la nostra storia, è la nostra tradizione, è la nostra identità e, allo stesso tempo, è un momento di rilancio dell'economia del nostro Paese, per i consumi

ma non deprimere l'economia del Paese. Dobbiamo farlo con responsabilità, con coraggio, ma senza battere in ritirata. Quindi ci sono la salute da un lato e l'economia dall'altro. Allo stesso tempo serve equilibrio nel momento in cui proroghiamo, immagino per oggettivi motivi sanitari, lo stato di emergenza. Occorre una maggior attenzione verso le imprese e le famiglie. Chiediamo quindi, signor presidente Draghi, più coraggio nel combattere l'aumento delle bollette dell'energia elettrica e del gas, più forza nel combattere l'aumento delle tasse e soprattutto più convinzione nel favorire la pace fiscale. Questo è il momento in cui dobbiamo andare incontro ancora di più alle famiglie e alle imprese. Ciò significa procrastinare la scadenza delle nuove cartelle, portare al 2022 la scadenza della rottamazione *ter* e del saldo e stralcio che sono andati in scadenza proprio ieri.

vivi da noi, quindi bisogna impedire che ci siano queste partenze illegali, e se riusciamo a tutelare la loro dignità, con un'integrazione reale

il Consiglio europeo del 16 dicembre dovrà esaminare lo stato attuale, considerando *in primis* gli sviluppi relativi al Covid-19 e la comparsa di questa nuova variante, che è un tema prioritario per la tutela della salute dei cittadini, ma è anche un tema interconnesso alla crisi globale e alla gestione della resilienza. Non a caso si parla, in questo momento storico, dell'era dell'antropocene o dell'era della resilienza: noi stessi abbiamo chiamato il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta dunque della capacità di resistere alle sfide e ai cambiamenti e farvi fronte, evitando di subire danni gravi e irreversibili, sia sul fronte ecologico e ambientale che su quello sociale ed economico. La pandemia ci ha dimostrato che le crisi assumono un carattere sempre più complesso e non si fermano alle frontiere, ma prima ancora del Covid-19 anche il cambiamento climatico e la diminuzione della biodiversità hanno dimostrato che i problemi sono globali e coinvolgono le comunità globali.

Tutti i *leader* devono confrontarsi per sostenere sforzi coordinati e per rafforzare quindi la nostra preparazione ad affrontare crisi future, direzionandola anche verso una visione sistemica e biocentrica e rafforzare la nostra capacità di risposta ai mutamenti e la nostra resilienza collettiva alle crisi che verranno. In futuro dobbiamo essere pronti a far fronte a crisi acute di natura diversa, che potrebbero anche essere molteplici, essere ibride, avere effetti a cascata o verificarsi simultaneamente, come già sta accadendo. presidente Draghi, il MoVimento 5 Stelle ha da sempre, nella propria storia, la missione di proteggere la casa comune e la comunità che vive in essa. Con il Governo Governo guidato dal presidente Giuseppe Conte abbiamo già affrontato l'inizio di questa crisi, in un momento in cui non c'era una valutazione del rischio, perché purtroppo non c'erano notizie sufficienti per poter supportare e capire quello che si doveva fare. Ci fa piacere che adesso questo Governo continui a fare bene e che ci sia unione anche qui all'interno. A volte resto un po' sconcertata, quando parlo con i ragazzi di Fridays for Future, con tutte le associazioni,

Per avere un simile modello economico, dobbiamo continuare a tutelare l'ambiente, il capitale naturale. So che in questo Consiglio parlerete dei servizi critici essenziali, da cui dipende la sussistenza dei cittadini: l'acqua, l'energia pulita, i trasporti sostenibili, il settore sanitario, le infrastrutture digitali, che il MoVimento 5 Stelle ha sempre portato avanti nelle sue battaglie. Il punto è che, se vogliamo affrontare gli effetti di questa crisi e di quelle che verranno, come l'aumento dei prezzi dell'energia, dei prezzi dell'energia, la scarsità delle materie prime, la sicurezza alimentare e la stessa crisi climatica (che è collegata alla migrazione), dobbiamo affrontarli con una gestione intersettoriale e transfrontaliera globale, non solo europea.

e che sicuramente tendiamo, come economia italiana, a tornare ai livelli di produzione pre-crisi entro la metà del 2022; queste sono le previsioni. andremo in questa direzione solo se al primo posto metteremo anche la tutela dell'ecosistema e del clima. In questi giorni il MoVimento 5 Stelle, come tutte le altre forze politiche, ha incontrato le associazioni ambientaliste italiane:

e per la loro competitività in un mercato globale, è giusto che forse ci sia una legge clima europea, una legge clima sovranazionale, perché è importante che che ci sia una armonizzazione fra i parametri del *carbon footprint* e tutto quello che verrà posto in essere. Concludo, Presidente, dicendo che noi noi possiamo tornare e sicuramente torneremo ad avere una vita migliore, perché alla fine un modello economico dovrebbe fare questo: tutelare la propria comunità in modo che possa vivere meglio,

degli organismi sovranazionali che possano gestire la crisi, perché purtroppo finora qualcosa non ha funzionato. Ho visto che si parla di un processo particolare per definire dei dispositivi integrati per la risposta politica alla crisi: ben vengano. Ma, oltre ai parametri economici, valutiamo anche i parametri ambientali e tuteliamo il nostro ambiente.

chi più chi meno, si usa finalmente questo termine. Vi è pertanto una soddisfazione abbastanza legittima, perché un grande maestro diceva che quando vedi le tue parole fiorire sulla bocca dell'avversario, qualcosa evidentemente sta succedendo. Al di là di questo, mi piace sottolineare che noi usiamo termini che enfatizzano un ragionamento politico, mentre in altre sedi, in altri schieramenti, si usano delle etichette. Noi di Fratelli d'Italia siamo i no vax più vaccinati del mondo; più vaccinati del mondo; siamo arrivati alla terza dose, siamo convintamente pro vax, però per qualcuno, evidentemente portatore di idee talmente deboli da non riuscire a confrontarle con le nostre,

il vaccino, infatti, salva il corpo ma non salva l'anima, quindi non è l'Eucaristia. In tutto questo, noi ci preoccupiamo di continuare a prospettare i nostri dubbi e le nostre perplessità.

Di queste 4,4 miliardi di dosi ne sono state consegnate quasi un miliardo.

della consapevolezza che bisogna vaccinare tutti per sconfiggere veramente il *virus*? L'Italia ha consegnato 134 milioni di dosi tramite il meccanismo Covax, come lei ha detto, e

cui veniva chiesto di rendere più trasparente il processo di ricerca, acquisto e distribuzione dei vaccini contro il Covid-19; ciò consentirebbe ai deputati, ma anche ai cittadini, di verificare in maniera più efficace le politiche dell'Unione sui vaccini. Dentro questi contratti, Presidente, secondo fonti giornalistiche, perché purtroppo non abbiamo a disposizione i contenuti di questi contratti e quindi ci dobbiamo attenere

a seconda della domanda. Il vaccino Moderna invece è il più caro di tutti, perché costa 18,80 euro a dose.

i segnalati, che mette a disposizione una cifra, calcolata in un miliardo di euro l'anno per i prossimi tre anni, per aumentare la dotazione del fondo per gli indennizzi

le segnalazioni registrate dalla Rete nazionale di farmacovigilanza dal 27 dicembre 2020 al 26 agosto 2021, quindi neanche tutto l'anno 2021,

Con il Covid, solo nel periodo dal 27 dicembre 2020 al 26 agosto 2021, sono state registrate 84.000 segnalazioni e i recettori di queste segnalazioni

queste segnalazioni in farmacovigilanza, Presidente, le faccio solo un esempio: è stata registrata un'incidenza anomala di miocarditi e pericarditi dopo i vaccini a mRNA. La necessità di segnalare immediatamente questi eventi è in rapporto stretto e diretto con la possibilità di trattare questi effetti, che sono assolutamente insignificanti se riconosciuti e trattati tempestivamente. Aifa ha

o evento avverso - come meglio si deve dire - è in particolare per i ragazzi sotto i trent'anni, ma la rete dei pediatri libera scelta non ha questa consapevolezza; questi sintomi che sono banali, se non trattati tempestivamente o

si fonda sulle esigenze di solidarietà sociale che impongono a una collettività di farsi carico dei danni che il cittadino abbia subito per essersi sottoposto ad una vaccinazione, anche nell'interesse della collettività. Sono le stesse parole che anche lei, signor Presidente, ha usato: ci si deve vaccinare per proteggere se stessi, i propri familiari e i propri colleghi colleghi di lavoro e la Corte costituzionale rispetto a questo si è pronunciata in modo assolutamente inequivocabile. Noi continuiamo a fare le solite domande e, al di

e di consapevolezza totali, per esempio attraverso i medici di medicina generale che, ad oggi, risultano essere coloro i quali in contumacia sono stati deputati ad effettuare il controllo dei loro pazienti e dei loro assistiti. Presidente, ci consenta un consiglio finale: prima di procedere alla vaccinazione dei bambini, arriviamo in tutti i modi a vaccinare quei 7 milioni di italiani, perché sono adulti e loro sì che si devono vaccinare. Il mondo non si può rovesciare: non possiamo vaccinare i bambini per proteggere gli adulti; dobbiamo finire di vaccinare gli adulti per proteggere anche i bambini. *(Applausi)*.

tra poco, in vista del prossimo Consiglio d'Europa, il Senato attribuirà al Presidente del Consiglio quella forza politica che in una democrazia rappresentativa può venire solo dalla volontà del Parlamento. Il suo intervento di poco fa, signor Presidente del Consiglio, è stato di grande spessore, non solo per i riferimenti alla corposa agenda del prossimo Consiglio d'Europa, a cominciare dalla lotta al Covid che l'Italia sta conducendo con grande attenzione e senso di responsabilità, ma, soprattutto, per l'idea di Europa che lei ha saputo disegnare a quest'Aula. Il prossimo Consiglio europeo è molto rilevante, anche per la delicatezza della fase che il mondo sta attraversando, perché il recente *summit* internazionale ha significativamente segnalato le preoccupanti minacce degli autoritarismi nei confronti delle democrazie le ultime gravi evidenze le abbiamo avute con le continue intossicazioni informatiche di molti processi elettorali democratici e con il piano eversivo contro l'elezione di Joe Biden. Oggi l'Europa è molto diversa dalla Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio del 1957; è più grande, più forte e più avanti nel processo di integrazione. Tuttavia, l'impresa non è ancora compiuta e manca l'ultimo miglio, il più difficile perché, mentre l'unione economica ha fatto importanti passi avanti, da decenni l'unione politica è in stallo per il conflitto dei diversi interessi delle Nazioni europee. anni dal Trattato di Roma l'Europa ha passato momenti positivi e momenti difficili e ancora oggi sta vivendo grande incertezze, per le difficoltà dei rapporti tra l'Europa orientale e quella occidentale e per la pressione militare russa nei confronti dei confini dell'Ucraina, che rappresenta la punta più grave di queste difficoltà, ma anche perché dal 1989 il vecchio ordine mondiale bipolare è svanito e da allora il mondo vive - ed è così tuttora - una disordinata fase di transizione. La simultaneità di tante crisi economiche, ambientali, sanitarie, sociali e militari non è dovuta al caso, ma al loro reciproco alimentarsi, perché c'è un legame tra la crisi sanitaria e quella economica, tra il riscaldamento del pianeta e le migrazioni, tra le nuove tecnologie e la crescita delle disuguaglianze, tra la sfida tra gli Stati Uniti e la Cina e le tensioni militari dell'indopacifica. In realtà, l'intero pianeta è sottoposto a forti instabilità e solo l'unità politica dell'Europa può dare agli europei la possibilità di contare nel mondo. il completamento del cammino verso un'Europa più solidale, più unita, più forte può essere ripreso. Il presidente Draghi ha parlato di bussola strategica. Noi possiamo anche osservare che nel nucleo centrale dei Paesi fondatori cresce la consapevolezza che i grandi problemi del continente non possono essere risolti senza una vera unità politica. Nel mondo, l'Europa gode del prestigio della sua storia, della sua cultura e dei suoi valori, ma la sua influenza sugli equilibri del pianeta e sui processi di pace è sostanzialmente irrilevante. Questo è il punto: il *deficit* dell'Europa è istituzionale e politico. Non è una federazione né una confederazione, ma un'unione di Stati tenuti insieme da trattati. Non ha una Costituzione ed è retta da un sistema sostanzialmente intergovernativo, che può decidere solo all'unanimità dei 27 Paesi membri. la paralisi, molto rischiosa, di una gestione non coordinata delle migrazioni e il grave ritardo in politica estera e di difesa. Negli ultimi decenni i pericoli per la pace si sono moltiplicati e saremmo molto miopi se pensassimo che per l'Europa sia sufficiente volere la pace per averla. Oggi, nel confronto geopolitico, solo le grandi potenze continentali hanno voce in capitolo. Come lei ha sottolineato, presidente Draghi, un'Europa più forte e più integrata rafforza l'alleanza Atlantica e la rende più solida. Sappiamo che la priorità strategica degli Stati Uniti è passata dall'Atlantico al Pacifico e che c'è un punto di continuità tra le amministrazioni democratiche e repubblicane. Obama, Trump, Biden hanno preso atto che gli americani non sono più disposti a mandare i loro figli a morire in guerre che non considerano le loro guerre. Ad una situazione a così alto rischio l'Europa giunge senza un vero governo che, in suo nome, possa democraticamente decidere la politica estera e di difesa. Per l'Europa affrontare questi temi presuppone la capacità di aggiornare i trattati e sciogliere nodi sempre considerati divisivi. Nessuna politica estera e di difesa; nessuna difesa dalle atrocità nei confronti dei migranti, di cui ha parlato poco fa la senatrice Bonino, può coesistere con l'obbligo di decidere all'unanimità. Ugualmente, una vera unione politica presuppone un Parlamento europeo con più forza e che ci sia più chiarezza nel rapporto tra Parlamento, Commissione e Consiglio d'Europa. Infine, le tante contrapposizioni tra blocchi di Stati ripropongono con forza un'Europa a più velocità. Signor Presidente del Consiglio, come le ho già accennato, ho molto apprezzato la visione dell'Europa che lei ha espresso poco fa nel suo intervento. Non avrei mai, però, affrontato questi temi, se, in occasione della firma dell'intesa tra l'Italia e la Francia, non l'avessi sentita affermare, a proposito dell'Europa: «il «il senso più profondo di questo trattato è che la nostra sovranità, intesa come la nostra capacità di indirizzare il futuro, può rafforzarsi solo attraverso una gestione condivisa delle sfide comuni»; e neanche

è stata pronunciata da lei, presidente Draghi, e da Macron: sovranità, sovranità europea. L'avete fatto in perfetta sintonia con il cancelliere Scholz, la cui coalizione ha sottoscritto un accordo di Governo che prevede prevede - non l'avevo mai sentito in un accordo di Governo di questa Europa - uno Stato federale europeo, una difesa europea e la fine dell'unanimità. Presidente Draghi, i suoi ideali europei autorizzano il Senato a invitarla a porre ai suoi colleghi del Consiglio europeo, assieme a Macron e Sholtz, il tema della sovranità europea, così come lo ha posto pochi giorni fa mentre firmava il trattato con la Francia. Lei può farlo; anzi, deve farlo, sapendo che l'obiettivo è ambizioso, che il cammino difficile e che le incognite politiche sono numerose, ma anche sapendo che, se l'Europa non è capace di andare avanti verso il traguardo passo dopo passo, non arriverà mai.

Immagino che sia piuttosto provato per aver dovuto ascoltare da questa mattina una sequenza significativa di sollecitazioni da parte dei parlamentari, come peraltro è suo dovere fare. scuso in anticipo se anch'io aggiungerò alcune ripetizioni ascoltate in questo dibattito. In pochi minuti ci tenevo a fare alcune sottolineature in relazione al contenuto del prossimo Consiglio europeo rispetto al quale lei avrà la responsabilità

grazie a tutti una fase molto difficile, però, come abbiamo fatto tutti, anche i colleghi presenti in quest'Aula, essendo stati destinatari della somministrazione di un vaccino, abbiamo provato e toccato con mano

arrivati quasi a 100 milioni di somministrazioni soltanto in Italia in un panorama europeo che ne conta sostanzialmente 300 milioni. Questo miracolo e questa operazione sono stati possibili grazie a questa capacità che abbiamo saputo mettere in campo grazie a quelli che spesso chiamiamo medici e infermieri. Forse dovremmo precisare che quei medici e quegli infermieri spesso sono dottoresse e infermiere, così come donne erano le commesse dei supermercati, le insegnanti,

autodeterminazione dei singoli e un principio di libertà, che naturalmente è sacrosanto, con un principio di cautela, che per fortuna, Presidente, abbiamo saputo tenere fermo. Il principio di cautela è quello che ci ha consentito di tenere la barra dritta proprio sul terreno delle misure di sicurezza e che oggi ci fa dire che l'Italia ha raggiunto traguardi molto più positivi di quelli raggiunti dagli altri Paesi. Lo dico, signor Presidente del Consiglio, pensando anche a un'altra discussione che voi Capi di Governo avete la responsabilità di portare in seno al Consiglio europeo: il rischio di un cortocircuito tra il fatto che alcuni regimi democratici, che fino in fondo liberali non sono e che sono dentro il perimetro dell'Unione europea,

un rischio che peraltro ci mette nell'urgenza di esprimere il massimo della solidarietà a una grande professionista, una giornalista come Lucia Goracci, che è stata destinataria di una vicenda surreale in un Paese che sta dentro il perimetro dell'Unione europea. Questo non è ammissibile lei come Capo del Governo italiano ha la responsabilità di portare anche in seno alla discussione nel Consiglio europeo esattamente questo aspetto: il terreno della qualità delle democrazie presenti oggi nel perimetro dell'Unione europea. Questo vale per la Romania

contro il caro bollette, ancorché si tratti di misure congiunturali. È positiva questa suggestione, che però va tradotta in politiche concrete, in relazione al tema dello stoccaggio integrato delle scorte strategiche di gas, che danno il senso di una misura minimamente più strutturale. Ma c'è poco da fare e lei per fortuna lo ha citato nel suo intervento: o noi scriviamo a caratteri cubitali dentro le agende politiche dei Paesi e dell'Unione europea la parola decarbonizzazione oppure non ne usciamo; o noi consentiamo che la transizione ecologica sia la più rapida possibile e facciamo in modo che i costi che inevitabilmente produce non siano scaricati sulle fasce più deboli, oppure quella transizione - per citare un profeta dell'ecologismo di questo Paese - semplicemente non sarà socialmente desiderabile, e quindi non sarà e non potrà dispiegare i suoi effetti positivi. Termino Siamo alla vigilia di uno sciopero generale io penso che le istituzioni, la politica e partiti di ogni estrazione non debbano più ammettere, come è stato in qualche modo ammesso in parte in questa fase del dibattito pubblico, che si stigmatizzi l'utilizzo di un istituto che resta costituzionalmente previsto come è quello dello sciopero, nel segno del rispetto dell'autonomia dei sindacati. Semmai il nostro tema, come Governo, come politica e come Parlamento è farci carico delle

dobbiamo assumere questa responsabilità nei confronti di chi oggi rischia di pagare prezzi più alti di altri, perché c'è una segmentazione e il rischio di un allargamento della forbice della disuguaglianza che questo Paese non può permettersi. È pertanto nostra responsabilità dare non solo voce a quel disagio, ma abbozzare alcune risposte più efficaci di quelle che abbiamo messo in campo, a partire attualmente della prossima legge di bilancio. La ringrazio per l'attenzione, signor Presidente del Consiglio,

Signor Presidente, colleghi, presidente Draghi, come sappiamo, il prossimo Consiglio europeo avrà, ancora una volta, al centro dell'agenda politica il contrasto alla pandemia. La battaglia contro il virus non è ancora finita e in quest'ottica sarà fondamentale rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri. Al momento l'unica arma che si è rivelata efficace contro il Covid-19 è il vaccino; per questo il prossimo Consiglio il prossimo Consiglio sarà l'occasione per esigere da parte degli Stati membri l'impegno a estendere il più possibile la vaccinazione alla loro popolazione. L'Italia ha raggiunto un'ottima copertura vaccinale, e di questo ringrazio lei, Presidente, il generale Figliuolo e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato; ma non viviamo in una bolla. Il virus non conosce confini, è essenziale far sì che il resto dell'Unione e del mondo accelerino sull'immunizzazione per consentire che si arrivi a una copertura globale del 70 per cento come già concordato al vertice G20. Nell'Europa dell'Est la copertura vaccinale è scarsa; in quattro Stati la percentuale dei vaccinati con doppia dose è inferiore al 50 per cento. Parlo di Croazia, Slovacchia, Romania e Bulgaria. È necessario un maggiore impegno anche nei confronti dei Paesi africani, dove solo il 6 per cento della popolazione è immunizzato e dove nuove varianti potrebbero emergere rendendo meno efficaci i vaccini. il virus non ha colpito solo la salute delle persone, ma anche l'economia. Per questo bisogna mantenere alta l'attenzione sui prezzi dell'energia, lavorando affinché si riducano i costi per famiglie e imprese. Il *green deal* è certamente il futuro, ma intanto c'è un presente fatto di difficoltà, ed è a queste che bisogna dare risposte nell'immediato. Il Governo, come Forza Italia ha chiesto, ha stanziato una cifra ragguardevole per limitare gli effetti del caro bollette, ma siamo d'accordo con lei, presidente Draghi, sul fatto che, se si rendesse necessario, si dovrà intervenire ulteriormente per rassicurare gli italiani. Occorre proseguire nel cammino verso la transizione energetica, ma allo stesso tempo impegnarsi affinché questa sia più sostenibile. Il percorso verso un'Europa più *green* non deve consumarsi sulla pelle di lavoratori e imprese; la transizione *green* deve essere senz'altro un obiettivo, ma non può diventare un'ideologia. Massima attenzione andrà rivolta anche al settore dell'*automotive*, fiore all'occhiello dell'economia italiana. L'obiettivo di eliminare le auto diesel e a benzina entro il 2035, per esempio, rappresenta un traguardo ambizioso che incontrerà diversi ostacoli. Per questo si dovranno accompagnare e sostenere le aziende del settore nella loro riconversione. In questo contesto, poi, dovrà essere rivolta massima attenzione al ruolo ancora più decisivo che potrà rivestire la Cina. Non è un mistero che Pechino detenga gran parte delle preziose riserve minerarie necessarie alla transizione ecologica. Diventare ancora più dipendenti da un regime illiberale come quello cinese, Presidente, sicuramente suscita in noi forte preoccupazione. C'è poi il tema del nucleare di quarta generazione, su cui tanto si sta discutendo a livello europeo e su cui anche l'Italia dovrebbe riflettere e aprire un confronto costruttivo, senza pregiudizi ideologici né preclusioni. Oggi dal commissario Timmermans abbiamo appreso della marcia indietro relativa alla proposta di direttiva sulla *performance* energetica degli edifici, che avrebbe impedito la vendita delle case non rispettose di determinati *standard* energetici. Forza Italia ne è soddisfatta, dal momento che avevamo espresso grande preoccupazione al riguardo. Il commissario europeo sembra anche sdoganare il superbonus italiano per le ristrutturazioni, per cui ne approfitto, presidente Draghi, visto che si avvicina l'approvazione del disegno di legge di bilancio, per chiederle il rinnovo di tale misura anche per le case unifamiliari a prescindere dal reddito; per non interrompere gli effetti positivi sull'economia ottenuti grazie a questa misura che, oltretutto, contribuisce in modo determinante al risparmio energetico. La transizione ecologica non può essere il mezzo per arrivare a una decrescita felice, ma dovrà essere l'occasione per aprire nuove strade e nuovi scenari imprenditoriali grazie a tecnologie all'avanguardia, in armonia con l'ambiente. Per quanto riguarda i fenomeni migratori, molti dubbi pone, Presidente, la riforma di Schengen che penalizza ancora l'Italia rendendo più facili i respingimenti verso gli Stati di primo approdo, compreso il nostro naturalmente. Come ho più volte ricordato in quest'Aula, il nostro Paese deve impegnarsi con maggiore vigore a riformare il Trattato di Dublino, superando il principio del Paese di primo sbarco, per affermare quello per cui i confini Sud dell'Unione non sono né italiani, né greci, né spagnoli, ma sono confini europei e, come tali, vanno considerati. La strada maestra per gestire i flussi deve restare quella di una redistribuzione equilibrata. Ciò fermo restando che va rafforzato il cammino di cooperazione con l'Africa per sostenere concretamente lo sviluppo economico, rimuovendo così le cause profonde dei flussi migratori da quel continente. Come lo ha ben definito Papa Benedetto XVI, dobbiamo garantire il diritto a non emigrare, a essere messi cioè nelle condizioni di rimanere nella propria terra. C'è poi il delicato tema dei rapporti con la Russia. È evidente la necessità di richiamare la Federazione russa a ridurre le tensioni militari alla frontiera con l'Ucraina e nel far questo è fondamentale, da un lato, riaffermare il pieno supporto europeo all'integrità territoriale dell'Ucraina, ma, dall'altro, e siamo d'accordo con lei, Presidente, proseguire nel dialogo per evitare un'*escalation* pericolosa delle tensioni. Riallacciandomi inoltre a quanto detto dalla senatrice Bonino, l'identità dell'Unione europea si fonda su valori comuni che hanno radici cristiane, illuministe, greche e romane. In nome di queste radici non fatico ad affermare che le immagini che arrivano dal confine tra Polonia e Bielorussia inammissibile che si lascino soffrire dei bambini al gelo e nella neve per ragioni geopolitiche. Il regime bielorusso arresta gli oppositori politici, non garantisce diritti e libertà e sta portando la popolazione allo stremo. Non lasciamo sola quella gente. L'Unione europea si faccia sentire con maggior vigore. Il prossimo Consiglio europeo sarà anche l'occasione per discutere di difesa e del primo nucleo di esercito comune da dispiegare in situazioni di crisi. Forza Italia auspica la formazione di una simile realtà da tempo affinché l'Unione possa contare su una reale politica estera per rivestire un ruolo più importante a livello internazionale e affrontare al meglio le nuove sfide che le si prospettano. ragione ci auguriamo che si arrivi a questo nuovo traguardo il prima possibile. Per concludere, Presidente, mi auguro possa fare tesoro di questa giornata di confronto con il Parlamento italiano e che porti le nostre istanze in Europa. Forza Italia le augura naturalmente un buon lavoro e un buon Natale. *(Applausi)*.

Siamo contentissimi di ogni investimento nel sistema difesa e sicurezza del nostro Paese e dell'Europa di fronte alle minacce e ad una situazione geopolitica che definire fluida è un eufemismo. Ma ci sono dei "però". Trovo quantomeno interessante e curioso che il perseguimento di una strategia comune europea e, quindi, obiettivi comuni tra i vari *partner*, venga praticato attraverso la proposta di superamento del principio di unanimità. Quale maggioranza - mi domando io - deciderà quali sono gli interessi dell'Italia, per esempio? Perché questo vuol dire superare il principio di unanimità; la maggioranza vince. Non stiamo però parlando di un Paese che passa alla democrazia, ma di un accordo tra Paesi e il superamento del principio di unanimità è un salto nel buio laddove non venga definito esattamente infatti il diritto di decidere è il più forte in un sistema fra Paesi, secondo l'interpretazione realista del diritto internazionale e delle relazioni internazionali. Questo mi lascia molti dubbi. Una soluzione potrebbe essere quella la funzione fondamentale del rapporto transatlantico Stati Uniti, Europa, NATO. Ben venga un'unità della difesa europea e della politica estera europea laddove l'Unione europea non sia semplicemente interoperabile con la NATO, ma sia parte di essa, con una NATO che detta le priorità geopolitiche, considerando il fatto che tanto la NATO, quanto molti *partner* europei, hanno interessi che travalicano i confini d'Europa. E per quanto riguarda potenze come l'Italia e i Paesi dell'Est, spesso subiamo minacce diverse. Di conseguenza c'è bisogno di un ombrello, di un'alleanza che tutt'altro che morta - né cerebralmente, né fisicamente - necessita semplicemente di essere utilizzata per come è nata, cioè come un'alleanza militare. Ci sarebbe altro da dire, ma non ne ho il tempo. Passo quindi al tema delle migrazioni. Ieri c'è stata la riunione settimanale del Collegio dei commissari europei, che a proposito ha fatto due osservazioni. La prima riguarda la modifica del codice Schengen a tutela dei Paesi che subiscono i movimenti secondari. È interessante. Con movimenti secondari - lo sappiamo tutti - si intende riferirsi ai migranti che dal Paese di primo approdo si spostano verso altri Paesi europei.

Il problema della migrazione è un problema europeo, non può essere un problema di alcuni Paesi europei: l'Italia è forse la *bad* *company* dell'immigrazione d'Europa? Tra soci, in una società, si dividono utili e perdite, di conseguenza questo mi stupisce e mi amareggia, soprattutto in un contesto come questo Parlamento in cui si parla di Europa come di un ideale fantastico. La seconda parte del tema migrazione ricade in un altro sistema, con il problema alle porte d'Europa, in Bielorussia. È chiaro che quello, però, non è più un problema di migrazione economica e climatica,

però, non è una novità: la Turchia qualche anno fa ha incassato sei miliardi di euro dall'Europa per non utilizzare i flussi a nostro svantaggio e a nostro detrimento, in particolare a detrimento dei Paesi dell'Europa centrale. Di conseguenza, non ci stupiamo del fatto che l'immigrazione non sia un problema di politica interna, ma un problema di difesa e sicurezza estera ed è questo che dobbiamo tenere presente: una nuova generazione di arma utilizzata contro di noi. di noi. Parliamo dell'Ucraina e della Bielorussia, ma dobbiamo parlare della Russia, perché è innegabile che, così come i migranti al confine polacco-lituano sono uno strumento di pressione della Russia verso l'Europa, allo stesso modo l'esercito russo alle porte dell'Ucraina è uno strumento di pressione politica verso di noi. Abbiamo due considerazioni da fare in proposito. L'equilibrio economico-energetico tra Russia ed Europa è in questi termini: nel 2019 l'Europa aveva un fabbisogno di 500 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il cui 39 per cento circa veniva dalla Russia. La Russia però - dobbiamo ragionare anche dal suo punto di vista - ha il 20 per cento del PIL realizzato tramite l'esportazione di materie prime energetiche verso l'Unione europea. è biunivoco, non sono solo loro che fanno pressione su di noi, anche noi possiamo fare pressione su di loro. Certo è che se le capacità di stoccaggio d'Europa sono un quinto del fabbisogno, è difficile accumulare riserve per poi farle scattare nel momento giusto. A questo proposito, dico anche che una posizione estrema sull'allineamento strategico dell'Ucraina è pericolosa. In questo momento, l'Europa preme per un'Ucraina all'interno dell'Unione europea e questo è estremamente pericoloso, perché determina una polemica con la Russia, che potrebbe allinearsi con la Cina e nell'Indo-Pacifico è uno scenario di cui neanche parlo perché non ne ho più il tempo. L'ultimo argomento il vertice con l'Organizzazione per l'unità africana. Sottolineo che per la transizione ecologica avremo bisogno di quelle materie prime di cui è ricca l'Africa e sulle quali sta mettendo le mani la Cina (cito solo il cobalto in Congo). Per la transizione ecologica non è solo una questione di gas e di nucleare, ma di materie prime per sostenere il passaggio alle fonti rinnovabili.

cosa ci ha insegnato questa crisi? Il Covid non ha fatto altro che far esplodere le contraddizioni che già esistevano prima della crisi.

per non parlare del settore del digitale, dove la potenza di fuoco dei giganti statunitensi e cinesi ha messo chiaramente in mostra l'arretratezza dell'Unione europea. Questo è davanti agli occhi di tutti, ma la crisi globale ne ha resi evidenti e ne ha accelerato gli effetti. del Consiglio, vorrei partire da queste premesse, per inquadrare il contesto attuale. Domani dovrete parlare di resilienza, energia e sicurezza. Per affrontare le sfide che abbiamo davanti, abbiamo bisogno di un modello che sia in discontinuità con quello dell'era pre-pandemica.

Ministro. Le chiediamo dunque di avere la forza e il coraggio per prendere in mano l'Unione e per fare quello che altri non sono riusciti a fare: cambiare la struttura dell'Unione Ad esempio, le chiediamo di attuare quanto scritto nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, quando si parla di piena occupazione e - perché no? - inserirlo o spingere per inserirlo nello Statuto

perché non cambiare le parole e dire che è un'economia eco-sociale di mercato, fortemente competitiva nei confronti dei Paesi *extra* UE. Chi può farlo, signor Presidente del un filosofo statunitense di fine Ottocento, che si chiamava John Dewey, diceva che il bisogno più sentito della natura umana è quello di sentirsi e di essere importanti. Lei ha già vissuto questa fase umana, quando salvò l'euro e fu al centro delle attenzioni di tutto il mondo. Quindi lei ha di fronte la possibilità di fare quello che altri non hanno fatto, anzi di riuscire dove altri hanno fallito. È il momento di prendere in mano le redini dell'Europa e provare a cambiarla profondamente, non a parole, ma con i fatti. La domanda è se lei ne ha la voglia, se ne ha l'intenzione e se ne ha la determinazione. cambiare l'Europa per avere un maggiore livello di capacità interna, in termini di produzione di energia, di sicurezza informatica, di capacità di gestione e utilizzo dei dati, nonché un aumento della resilienza agli *shock* asimmetrici che avvengono in altre parti del mondo. Per fare tutto questo bisogna superare il concetto di competizione intracomunitaria e lavorare in cooperazione tra gli Stati e tra gli attori industriali dell'Unione europea. La ricchezza prodotta deve essere poi redistribuita, a beneficio dei cittadini dell'Unione europea. La trasformazione deve avere una visione ecologica, per fare in modo che l'Unione sia un campione mondiale da questo punto di vista. Questo è il senso delle proposte che abbiamo fatto prima e che il MoVimento 5 Stelle ha presentato in una mozione, che abbiamo presentato all'Assemblea nel marzo di quest'anno. La competizione interna all'Unione non ci porta a essere un competitore forte, ma abbiamo bisogno di cooperazione. Prima il senatore Zanda parlava della Comunità europea, usando una parola bellissima, per per avere una competizione reale con i grandi giganti, con i grandi attori mondiali come gli Stati Uniti e la Cina - con gli Stati Uniti per il mondo del digitale e con la Cina dal punto di vista del percorso industriale e per cominciare quindi ad intraprendere sul serio e con forza un percorso che vada verso l'autonomia strategica. Solo due temi. Sulla sicurezza informatica ricordiamoci che le principali dorsali paneuropee di fibra ottica sono in mano a società o a fondi statunitensi e che sul tema del *cloud* le più grandi società sono tutte statunitensi, anche se i cinesi non si fanno mancare ovviamente di avere delle *region* in Europa. Il progetto Gaia X, che parla del *cloud*, è un progetto *cloud*, è un progetto debole, perché è una federazione e in questa federazione ci sono anche i grandi attori statunitensi e cinesi; noi invece avremmo bisogno di una cosa diversa, avremmo bisogno di un qualcosa come il vecchio progetto Airbus, in cui c'era un consorzio di imprese europee che affrontavano il sistema. Oggi Airbus è il più è il più grande competitore al mondo dell'americana Boeing. Dal punto di vista industriale, l'asimmetria ci ha fatto vedere come l'Italia sia un grande produttore e fornitore di pezzi di qualità ma questo si regge anche sul fatto che i salari in Italia negli ultimi trent'anni, come sa, non sono aumentati, anzi sono diminuiti, a differenza di tutti gli altri Paesi dell'Europa. E allora abbiamo bisogno di un cambio di passo. Le faccio un esempio, una cosa che sembra di dettaglio; le parlo dei magneti permanenti. I magneti permanenti sono alla base della transizione ecologica: servono per fare le turbine eoliche e per l'industria dell'*automotive*. L'Europa importa il 95 per cento dei magneti permanenti dalla Cina, che è il produttore mondiale più forte con il 95 per cento della produzione mondiale. Dobbiamo produrre i magneti permanenti, permanenti, ma, per fare questo, dobbiamo superare un *gap* sulle sostanze di base; in particolare ne potremmo citare una, il neodimio, che è una terra rara. Ma le terre rare l'Europa le importa per il 100 capire che il progetto ERMA, che è l'alleanza europea per le materie prime, deve essere spinto con forza. Un'industria del futuro, che è un'industria ecologica, un'industria profonda, dove lavoriamo sul tema del digitale, non può essere disgiunta dalla possibilità di superare questo *gap*, che è un *gap* tutto europeo. Forse dovremmo pensare a fare una cosa che potremmo chiamare "miniera nazionale", cioè una grande fabbrica che, partendo dai RAEE, produca quelle terre rare e quegli elementi, come il litio, che sono alla base delle batterie e quindi degli stoccaggi dell'industria dell'*automotive*, che servono a far cambiare il sistema. Forse dovremmo fare questo. Ecco, quando parliamo di sicurezza, resilienza ed energia pulita, dovremmo fare queste cose; però queste cose prevedono una grande cooperazione tra Stati. può e deve onorare il mandato che il Parlamento le ha dato. Lei deve essere la testa d'ariete nella trasformazione dell'Unione. È questo il vero compito che le abbiamo assegnato. Lo faccia e dimostrerà che la scelta di individuarla come Presidente del Consiglio ha avuto un senso, che travalica le logiche nazionali. Lo faccia e avrà il plauso dei cittadini che vogliono un'Europa che sia vicina al popolo e non vicina alla finanza o a logiche di *business* che sono invece lontane dai loro bisogni. Lo faccia, Presidente, lo faccia.

dalla senatrice Granato, n. 2, dai senatori Stefano, Lorefice, Candiani, Giammanco, Bonino, Nannicini, Garavini, Steger e De Petris, n. 3, dal senatore Ciriani e da altri senatori, e n. 4, dal senatore Paragone e da altri

Signor Presidente, intanto volevo ringraziarvi per tutti gli spunti e per i complimenti che molti di voi hanno fatto all'azione di Governo. Vorrei fare due osservazioni di carattere generale. è che questo Governo, come avete visto, affronta il cambiamento non con spirito difensivo, ma con coraggio e con determinazione. Di questo credo che tutti voi abbiate dato atto. Ma è anche, devo dire, un cambiamento molto difficile. Pensate che nell'arco di due anni e mezzo o tre anni è cambiata la nostra prospettiva in maniera radicale: il Covid, la transizione ecologica, la transizione digitale, la necessità, le nuove sfide geopolitiche. È un periodo di grandissimo cambiamento e questo suggerisce l'altra l'altra linea dominante dell'azione di Governo. Il cambiamento va sì affrontato con coraggio, se volete con lungimiranza e intelligenza, ma costante in questo deve essere lo sguardo ai più deboli, altrimenti il cambiamento non avviene La seconda considerazione di carattere generale, che però in un certo senso risponde a un punto che molti di voi hanno sollevato, riguarda i vaccini e l'azione del Governo nella campagna vaccinale. A questo proposito, prima di tutto desidero porgere un ringraziamento pubblico al generale Figliuolo come alcuni di voi hanno osservato - lo sforzo organizzativo e logistico è stato imponente. nelle varie posizioni che si possono prendere al riguardo, vorrei soltanto ricordare che noi ci siamo ripresi una normalità, con la quale possiamo guardare a questo Natale e alle feste

Ora vengo a dei punti sollevati da alcuni di voi. Condivido col senatore Renzi il senso straziante delle parole del professore di storia Carmina. È una lettera bellissima quella che scrive ai suoi studenti e va ricordata per sempre.

pensare a un ritorno del Patto di stabilità nella sua formulazione Quanto è realistico oggi pensare a una riformulazione del Patto di stabilità nei termini in cui è stato in vigore fino a poco prima della pandemia? Secondo me, non è realistico. Le regole del Patto di stabilità si sono dimostrate inefficaci e procicliche, cioè dannose.

considerare l'avvento della pandemia, le enormi spese che abbiamo dovuto affrontare per la pandemia stessa, ma soprattutto le enormi spese che dovremo affrontare per vincere quelle transizioni a cui l'Unione europea ci chiama: la transizione ecologica, la transizione digitale e poi la difesa. Mi riferisco a queste regole nella loro formulazione di allora insieme ad altre regole, come anche a quella sugli aiuti di Stato. Come si può pensare di fare una transizione ecologica o una transizione digitale senza un ruolo attivo senza un ruolo attivo dello Stato nel processo di creazione delle nuove imprese? Quindi, credo che lo sforzo di riflessione a cui si appresta tutta l'Unione europea sarà profondo e complesso. Peraltro, la Commissione ne è consapevole;

perché quel che ho appena detto è in effetti quello che sta succedendo in tutto il resto d'Europa. È molto difficile tornare al passato. Detto questo, voglio però aggiungere che le regole servono

cioè la creazione di un bilancio comune, sia nel creare solidarietà per affrontare come quelli che abbiamo vissuto, sia nel creare in prospettiva quella che viene definita una capacità fiscale, che permetta ai Paesi di affrontare la stabilizzazione del ciclo economico, in maniera tale da non aggravare la loro posizione quando ci sono crisi, com'è successo peraltro nel periodo successivo alla crisi finanziaria. Professor Monti, sono d'accordo con lei: si è rafforzata l'Italia in l'Europa, si è rafforzata l'Europa in Italia e si è rafforzata l'Italia nel mondo. Devo però aggiungere che la sensazione di ritrovata fiducia da parte del resto del mondo, da parte dell'Europa e dell'Italia porta anche a una grande responsabilità. Porta la responsabilità del Paese a dimostrare che questa fiducia è meritata.

che sono stati dati all'Italia, il che significa che gli altri Paesi europei hanno accettato di tassare i loro cittadini per dare soldi all'Italia.

dell'energia. Come ho detto prima, il Governo sta intervenendo in una misura che non ha precedenti per proteggere gli strati più deboli della popolazione,

con una cifra che, se ci pensiamo un momento, è di circa 8 miliardi in sei mesi;

Si pensa che nella seconda parte dell'anno i prezzi del gas potranno scendere - questo è quanto ci dicono le previsioni dei mercati - ma, come rilevavo, ci sono delle componenti strutturali che probabilmente renderanno questa discesa meno marcata di quanto sarebbe desiderabile, per cui dovremo forse rassegnarci a un aumento strutturale del prezzo dell'energia. impone dunque anche una riflessione di carattere strutturale su questo. La Commissione europea ha già fatto proposte per gli acquisti congiunti di stoccaggi, ma vi vi sono anche altre proposte: bisogna che le interconnessioni siano migliorate, in maniera tale da poter sovvenire ai vari Paesi dell'Unione europea con forniture provenienti da altri Paesi dell'Unione. il prezzo del gas verrà influenzato anche da fattori geopolitici. In particolare, il gasdotto Nord Stream 2 è o potrebbe divenire uno strumento negoziale nella politica tra l'Unione europea e la Russia. Se dovesse diventare parte dell'apparato sanzionatorio - noi ci auguriamo che non debba essere necessario - è chiaro che l'influenza sul prezzo del gas sarà molto marcata:

a fronte del sacrificio di tanti cittadini, ci sono degli enormi profitti realizzati da coloro che producono con

c'è il guadagno che deriva dal prezzo del gas e dalla possibilità di vendere l'energia a quel prezzo. Questo è uno schema di formazione del prezzo europeo.

chiaramente suggeriscono che è venuto il momento di una riflessione strutturale sulla questione.

in particolare, noi paghiamo probabilmente più di tutti gli altri Paesi: la Germania paga molto meno di noi; la Francia un po' più della Germania e un po' meno dell'Italia; la Spagna credo che sia più o meno a livello italiano.

la decisione di bloccare gli investimenti negli impianti a carbone, di bloccare le estrazioni e i finanziamenti degli impianti a carbone.

La senatrice Bonino ed altri hanno sollevato il problema dei diritti umani, del rispetto dei diritti umani al confine tra tra Russia e Polonia. Condivido completamente le osservazioni della senatrice Bonino. Tra l'altro, si tratta di 3.000-4.000 persone e noi, solo quest'anno, ne abbiamo prese più di 63.000. Quindi, neanche i numeri giustificano quei trattamenti inumani, e questo verrà detto al Consiglio europeo. Più generalmente, il problema è molto complesso. è molto complesso. È un discorso molto lungo e, quindi, non è il momento di affrontarlo. Posso, però, dire alcune cose. Il primo sforzo, forse, è quello di deideologizzare la questione della migrazione. Certi numeri non sono assolutamente sostenibili, certi altri sì. Come si fa a fare in modo che le migrazioni diventino risorse? Qui, purtroppo, abbiamo moltissimo da fare. Come italiani abbiamo moltissimo da fare, non per migliorare, ma per costruire un sistema di accoglienza che faccia diventare quelle persone delle risorse sul mercato del lavoro e, infine, degli amici degli italiani e non dei nemici. Se noi non non facciamo questo, produrremo solo dei nemici. E abbiamo già fatto questa discussione un'altra volta, ma ripeto che, con questo sistema di accoglienza, le capacità che l'Italia ha di assorbire le persone legalmente presenti in Italia sono poche. Quindi, dobbiamo investire molto di più e probabilmente ricostruire il nostro sistema. Perché, poi, parlo di deideologizzare la questione? Sento parlare di difesa delle radici e dell'identità. Ora, io non voglio entrare nella definizione di che cosa sono le radici e di cos'è l'identità. Ma credo che un modo di difendere le radici e l'identità sia sia quello di affermare e vivere i valori caratteristici delle nostre radici e della nostra identità. Per esempio, uno di questi valori è la solidarietà; un altro, però, è la responsabilità. Bisogna stare attenti - secondo me - a ragionare in termini possibilmente non ideologici, ma pragmatici sull'argomento.

Io ne sono convinto. Per affrontare sfide globali occorre andare oltre i confini nazionali. È chiaro e si è visto. La pandemia, l'ambiente, il cambiamento climatico, la difesa europea, la transizione digitale ed ecologica: sono tutte sfide che, per loro stessa definizione, travalicano i confini nazionali. Quindi, bisogna trovare un modo per lavorare insieme. senatrice L'Abbate ha richiamato la necessità che tutti facciano la loro transizione, che non ci siano Paesi che si tirano Qualche passo avanti è stato fatto durante il G20. Naturalmente, è un processo lungo, ma il fatto che sia lungo e difficile non ci esime dalla responsabilità del richiamare tutti quei Paesi a fare la loro transizione. Naturalmente - come dicevo prima - le condizioni di partenza sono diverse e la transizione non è immune da costi. Basta pensare, infatti, che il Paese che produce il 50 per cento dell'acciaio mondiale ha quasi tutti gli impianti a carbone. Ora li sta convertendo in impianti a gas e il prezzo del gas aumenta, e aumenta strutturalmente perché, se la transizione in quel Paese continua, l'aumento sarà strutturale. Senatore Zaffini, i numeri dell'Europa sono migliori o come quelli degli altri Paesi nel mondo. Il problema non è solo la non è solo la quantità di vaccini che si danno; oggi è molto più importante riuscire a somministrarli. Oggi la dimensione logistica è diventata la più pressante, tanto è vero che con tutte le donazioni i tassi di vaccinazione in Africa restano ancora molto bassi. Condivido l'analisi delle complessità attuali del senatore Zanda e la necessità di progredire verso l'unione politica. In effetti, oggi abbiamo discusso molte

Di fronte alle sfide che l'Europa si trova ad affrontare con l'unanimità noi non reagiamo. È stata una cosa meno sentita negli scorsi anni, quando l'ombrello protettivo dell'alleato atlantico ci aiutava a non affrontare queste sfide. Oggi le priorità geopolitiche del nostro alleato stanno modificandosi. Altre parti del mondo stanno acquistando acquistando più importanza e, quindi, ci dobbiamo attrezzare. E ci attrezziamo soltanto se riusciamo a decidere e, per fare ciò, bisogna superare l'unanimità. Ciò vale per la politica estera, per la politica della difesa e anche per altre sfide. la necessità di avere compiti chiari, ben definiti e decisioni rapide è essenziale. Qui viene il punto: forse non si riesce ad arrivare a quel punto senza un percorso convinto verso l'unione politica. Ci si chiedeva prima come si fa a non avere una decisione unanime e a rassegnarsi i miei figli vadano a combattere e a morire per decisione di un altro, perché c'è la maggioranza. Ci si riesce soltanto se ci avviamo convintamente verso un'unione politica, verso un'unione in cui tutti ci sentiamo membri dello stesso Stato.

Quando ricordiamo quanto successo durante gli ultimi mesi e diciamo che lo sforzo logistico - come ho appena detto - è stato imponente, in effetti dobbiamo ricordare il

dell'assistenza che è stata prestata a milioni di famiglie. Per quanto riguarda i sindacati, da parte del Governo non c'è stata alcuna volontà punitiva, tant'è che la settimana prossima - credo lunedì o martedì - abbiamo convocato la prima riunione per aprire un tavolo su una possibile riforma delle pensioni: c'è quindi volontà di colloquio, di condivisione, di ascolto, come abbiamo fatto peraltro sul decreto-legge sulla sicurezza sul lavoro.

L'impressione degli ultimi scambi che ci sono stati è che da parte della Russia

che c'è necessità di rimanere - come ho detto nel corso della telefonata con il presidente Biden - ingaggiato. Ciò significa

a non forzare le cose, a mantenere questo ingaggio e a pretendere, però, il rispetto degli accordi di Minsk da parte sia del presidente Putin che del presidente Zelensky.

cosa avviene per quanto riguarda gli spostamenti delle truppe al confine con il Donbass; cosa fa il presidente Zelensky a proposito del riconoscimento del Donbass; cosa fanno entrambi a proposito dello scambio di prigionieri.

a tutti i Ministri e Sottosegretari, gli auguri di buon Natale, a nome di tutta l'Assemblea del Senato.

Signor Presidente, se è vero che con il virus dovremo convivere ancora a lungo, dobbiamo puntare a migliorare costantemente le strategie di contrasto. La nuova ondata evidenzia che i Paesi europei, che non hanno seguito l'esempio italiano sul *green pass* anche nei luoghi di lavoro e sui tamponi a pagamento, oggi sono i più colpiti. Ma la nuova ondata sta dicendo anche che l'elemento più debole è la bassa omogeneità delle misure tra i Paesi europei. Oggi l'Europa chiede conto all'Italia delle decisioni sulle frontiere, ma forse dovrebbe interrogarsi sul perché, mentre l'Italia teneva alta teneva alta la guardia contro il virus, altrove si smantellava gran parte delle forme di prevenzione. Su questo si deve fare di più, non limitandosi più a una politica di raccordo, ma puntando a una maggiore omogeneità delle misure. Dobbiamo fare un passo in avanti sulla crisi energetica e sulle questioni geopolitiche collegate. Per questo, se è positivo il rafforzamento delle risorse contro il caro bollette per contrastare a monte l'aumento dei costi, bisogna, però, approvare velocemente in sede europea l'acquisto e lo stoccaggio collettivo di gas. Tuttavia, questa crisi presenta anche altre sfide: una famiglia italiana su sei è in una condizione di povertà energetica, che vuol dire non solo difficoltà a pagare le bollette, ma anche impossibilità a migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione con elettrodomestici di vecchia generazione e case meritevoli di ristrutturazione. C'è, poi, la partita più importante, quella per la decarbonizzazione di un Paese che ha condizioni ottimali per sfruttare le potenzialità delle rinnovabili. Servono su questo incentivi strutturali, ma anche interventi innovativi, come quelli per l'autoproduzione solare e per le comunità energetiche dove l'energia prodotta viene distribuita tra le famiglie più bisognose. Occorre, naturalmente, una decisa risposta a chi sta sfruttando il problema energetico e usa i migranti come indebito strumento di ricatto politico ai danni dell'Europa. Sempre su questo tema, se - da un lato - l'Italia non può essere lasciata sola - dall'altro - concordo con lei quando dice che serve un nuovo approccio con corridoi umanitari e quote di ingresso stabilite per una migrazione come opportunità. Paesi come la Svezia, la Germania e l'Austria, dove la percentuale di stranieri è decisamente più alta, ci dimostrano che i fenomeni migratori non sono solo una questione di sicurezza e di ordine pubblico. Non a caso, gli stranieri che sbarcano in Italia sperano di raggiungere proprio quelle Nazioni. Presidente Draghi, tra quarta ondata pandemica, turbolenze geopolitiche e necessità di proteggere la ripartenza economica, la lezione che se ne trae è sempre la stessa: le criticità del nostro tempo diventano minacce tutte le volte che l'Europa si divide. Vengono fronteggiate e addirittura si trasformano in opportunità per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo allorquando c'è l'unità di intenti tra gli Stati membri; una lezione, questa, che dovrà essere alla base della riscrittura delle regole comuni con più integrazione e - come dice anche lei - voto a maggioranza; ma anche trovando il giusto punto di equilibrio tra la solidarietà e il fatto che il debito che stiamo contraendo non venga lasciato in pegno alle future generazioni di europei. La fase che attraversiamo è delicata: richiede stabilità politica con un Governo che porti a termine il suo mandato, anche rispetto alle sfide del Piano Serve un'Europa che, nell'affrontare le sfide del presente, ponga le basi per il futuro, alimentando sempre di più il processo di integrazione.

grazie dell'attenzione che rivolge a questo Parlamento, presidente Draghi, anche nella misura in cui si impegna a rispondere in modo puntuale agli interventi dei singoli senatori. Gliene siamo molto riconoscenti, perché riteniamo che sia davvero un'attenzione, *in primis*, alle istituzioni e a questo Parlamento. Grazie! E grazie del fatto che una volta tanto l'Italia viene presa a modello e viene ammirata al suo interno e nel mondo per l'efficacia della campagna vaccinale e per l'obbligo di certificato verde, misure che stanno facendo scuola a livello internazionale. Anche l'ordinanza delle ultime ore che richiede il tampone ai vaccinati in arrivo in Italia va nella direzione giusta. È importante che essa venga concordata con l'Unione europea e comunicata bene, perché è il modo per garantire sicurezza senza di nuovo sospendere la mobilità all'interno dell'Unione. Bisogna poi continuare a insistere sulle vaccinazioni: un compito urgente se si pensa che il tasso medio di vaccinati in Europa è molto più basso che non in Italia, soltanto il 77 per cento degli adulti. Ciò vuol dire che un europeo su quattro continua a rappresentare un pericolo per sé e per gli altri. Ecco che serve ancora uno sforzo collettivo importante. Particolare attenzione da parte europea va data anche al potenziamento del programma Covax, perché non è immaginabile debellare il contagio a casa nostra se nel resto del mondo la pandemia continua a imperversare. Non a caso, l'ultima variante si è sviluppata proprio in Africa, cioè in quel continente che detiene il 17 per cento della popolazione mondiale, ma che finora ha avuto accesso solo al 3 per cento delle dosi di vaccino disponibili a livello globale. Ecco che bisogna potenziare gli aiuti affinché si proceda speditamente con le vaccinazioni anche nei Paesi extra UE. UE. All'ordine del giorno del Consiglio europeo, però, ci sono diverse tematiche spinose legate alla politica estera, a partire dalla situazione dei profughi al confine tra Bielorussia e Polonia. È palese che il regime bielorusso ha ingannato migliaia di profughi, reclutandoli in decine di villaggi in Siria, Iraq e Yemen, promettendo loro di entrare in Europa passando da Minsk. Al costo di migliaia di dollari a persona i profughi sono stati portati su voli nella capitale bielorussa; poi sono stati trasferiti alla frontiera con la Polonia con la promessa di oltrepassarla, per trovare magari lavoro in Germania o altrove; salvo poi venire usati come strumento di pressione contro l'Europa, lasciandoli al freddo e al loro destino davanti al filo spinato. Una strategia di questo tipo è disumana, usa i migranti nei confronti dell'Unione europea allo scopo di destabilizzarla. Ecco perché non possiamo tollerare un atteggiamento di questo tipo. Non è il caso di ritirare sanzioni verso la Bielorussia. È positivo che si sia posto fine ai voli in partenza dal Medio Oriente per la Bielorussia e che si stia cercando da parte europea di organizzare il rientro dei profughi nei rispettivi Paesi di origine, con tutte le difficoltà del caso. Non possiamo lasciare, che neonati e donne incinte muoiano assiderati dopo notti passate nei boschi, al freddo, nel tentativo di entrare in Europa. Lei ha ragione, presidente Draghi, bisogna provvedere alla creazione di corridoi umanitari europei, nonostante sia chiaro che l'operazione è orchestrata ad arte per mettere in difficoltà l'Europa; tutto ciò purtroppo, probabilmente, con l'avallo della Russia interessata, a sua volta, ad indebolire l'Unione, attraverso - ad esempio - le minacce militari all'Ucraina, ai confini della quale la Russia negli ultimi mesi ha più che raddoppiato il dispiegamento di proprie truppe. È un gioco pericoloso quello che sta giocando Mosca; può darsi che si tratti soltanto di un'azione intimidatoria volta a dissuadere Kiev dal voler entrare nella NATO, ma è sicuramente una mossa azzardata. Ecco perché è necessario che l'Europa chieda a Mosca di interrompere queste provocazioni. Mosca non può usare una minaccia inesistente come pretesto per creare una minaccia vera. Vogliamo una politica estera europea che si muova con sensibilità, ma anche con determinazione. Ecco perché riteniamo che, nel caso in cui non si riscontri alcuna *de escalation* da parte russa, si debbano adottare ulteriori sanzioni. C'è un'altra modalità che la Russia sta usando per mettere in ginocchio l'Europa: sta tagliando le forniture di gas per influenzare la politica internazionale, con il conseguente repentino aumento dei costi dell'energia. In Europa non si registravano bollette così alte da una decina di anni a questa parte. Ecco perché è molto positivo che l'Italia abbia richiesto la creazione di uno stoccaggio di riserve di gas e che sia intervenuta a livello nazionale con la forte riduzione dei costi. Allora, signor Presidente, ottima la bussola strategica; ottima l'insistenza da parte italiana sulla questione migratoria; ottimo l'intento di superare il veto all'unanimità; ottima la consapevolezza che necessitiamo di una radicale modifica del Patto di stabilità. Un invito, signor Presidente: porti al Consiglio europeo anche la necessità di non lasciare nel dimenticatoio la questione afgana. anche da parte nostra i più sinceri auguri di buon lavoro e di buone feste. *(Applausi)*.

Il fatto che l'attuale Presidente del Consiglio goda di un prestigio personale superiore a quello dei suoi predecessori degli ultimi anni è certamente un fatto positivo. Fratelli d'Italia le chiede di far pesare detto prestigio a favore degli italiani nelle varie questioni che verranno trattate, anche quando ciò potrà dispiacere a qualcuno dei nostri *partner* europei. Sulla questione pandemia e vaccini, ha parlato con la consueta competenza ed eloquenza il senatore Zaffini; voglio solo aggiungere l'esortazione ad evitare, nella corsa ad essere i primi nelle limitazioni, nei divieti e negli obblighi, di arrivare al punto di farci bacchettare dal vice Presidente della Commissione europea, come è successo oggi, quando Vera Jourova ha praticamente detto che siamo andati talmente avanti che rischiamo addirittura

Venendo al punto molto importante dell'agenda del Consiglio europeo, cioè la questione economica, il patto di stabilità è stato sospeso - sembra - fino al 2022. Questo vuol dire che fra un anno staremo discutendo - speriamo in modo più rispettoso del ruolo del Parlamento di quanto accade in questi giorni, in cui il Parlamento è praticamente escluso da una reale possibilità di incidere - una legge di bilancio per il 2023 sulla quale graverà il rischio di nuove misure di austerità, che potrebbero azzerare i risultati ottenuti finora, che comunque ci vedono ancora ben al di sotto del livello di prodotto interno lordo del 2019 e con un debito del 150 cioè 300 miliardi più di due anni fa, che graverà su di noi e sulle prossime generazioni; sempre che ci siano le prossime generazioni, perché questa è un'emergenza che non viene mai menzionata. Arriveremo quindi al totale del

quindi al totale del 150 per cento del rapporto-debito PIL, tenendo presente che dieci anni fa fu fatto cadere l'ultimo Governo del centrodestra guidato da Silvio Berlusconi perché eravamo arrivati all'insostenibile livello del 119

sia a lungo termine. Sappiamo infatti che queste politiche di austerità a suo tempo hanno fatto addirittura aumentare il debito, sappiamo che ci saranno delle resistenze da parte di Paesi che hanno, per un verso, un livello di debito più basso di quello italiano e, per un altro, la convenienza a tenere l'Italia in posizione di svantaggio, perché temono la concorrenza dell'Italia, delle sue aziende e dei suoi lavoratori. Le chiediamo - a proposito di economia - di difendere la specificità italiana sulla questione delle concessioni demaniali marittime, che oggi vede in pericolo centinaia di imprese e decine di migliaia di posti di lavoro. Strettamente connessa alla questione economica generale è la questione dell'energia, un altro punto dell'agenda del Consiglio europeo. È un punto particolarmente delicato, in un momento in cui il prezzo del petrolio è salito del 200 per cento e quello del gas del 30 per cento rispetto a due anni fa. Questo è un effetto del mercato. Ci sono, però, anche le politiche di transizione ecologica, che hanno dato un notevole contributo: il prezzo dei certificati, i cosiddetti permessi di emissione dell'anidride carbonica, che era sotto i 10 euro fino al 2018,

e delle aziende. Diventiamo così meno concorrenziali rispetto a chi, come la Cina e altri Paesi cosiddetti emergenti, non ha bisogno di alcun permesso per emettere anidride carbonica. Le ambiziosissime mete poste a livello europeo, anche con l'accordo dell'Italia, tra l'altro consentono al nostro Paese una quantità di emissioni che è del 28 per cento inferiore a quella della Germania, che pure ha le centrali nucleari, e forse anche su questo bisognerebbe lavorare. è soprattutto con la Cina e con gli altri Paesi cosiddetti emergenti. Il risultato sembra essere che le produzioni italiane si sposteranno in Cina, dalla quale compreremo prodotti, come i pannelli fotovoltaici, per ridurre le emissioni, ma quei pannelli saranno prodotti senza limiti di emissione. Pertanto il saldo rischia di essere: meno posti di lavoro e meno ricchezza prodotta in Italia,

e non quanto ci frutta magari una passeggera pacca sulla spalla nelle sedi internazionali e poi le spese le pagano le imprese, i lavoratori e le loro famiglie. Di certo siamo e saremo fermamente e duramente contrari a provvedimenti come

A noi la cosa pare preoccupante. Lei stesso ha detto che queste persone, se non le trattiamo abbastanza bene, diventeranno nostri nemici. La cosa ci preoccupa un tantino, anche perché si è pure verificato qualche caso di terroristi che sono arrivati in questo modo. L'Italia non ha firmato quella lettera di 12 Paesi dell'Unione europea che chiedeva aiuto all'Unione per gestire l'immigrazione, eventualmente anche con la disposizione di barriere di vario tipo. Lei stesso però, qualche giorno fa, ha detto che l'immigrazione è fuori controllo. Credo dunque che un ragionamento tra le due considerazioni vada fatto: non possiamo solo parlare di accoglienza e solidarietà, perché naturalmente chi arriva e ha diritto a stare qua deve essere trattato bene, ma non possiamo accogliere chiunque. il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha detto negli scorsi giorni che auspica un'Europa che sia un gigante politico e non un gigante burocratico. Un gigante però deve avere un cuore, dei principi e dei fondamenti, altrimenti è un gigante pericoloso.

passare per ambasciatore dell'Unione europea - pare non sia ambasciatore, ma è comunque un consulente del Parlamento europeo - che fa quelle foto vergognose, atteggiandosi a Vergine Maria con la barba. Dopo certe cose non stupiamoci se poi qualcuno non ha un sentimento immediatamente positivo nei confronti dell'Europa. Lei, signor Presidente, ha firmato la lettera durissima fatta da alcuni Capi di Governo contro la legge passata in Ungheria che vietava la distribuzione di materiale omosessuale o pornografico ai minori. Ebbene, ormai è fatta; ho parecchi dubbi però che quella legge sia contro i principi europei, dell'Europa di Adenauer, De Gasperi e Schumann. Ma allora, se questo è il problema, parliamo anche dei Paesi che consentono l'utero in affitto, che è una vergogna e una barbarie, in cui i bambini sono una merce e le donne un mezzo di produzione. Detto questo, ricambiamo gli auguri di buon Natale, nella speranza di un operoso lavoro in sede europea.

presidente Draghi e il sottosegretario agli affari europei Amendola andranno al Consiglio europeo con alle spalle la gran parte delle forze politiche che sostengono il Governo fornendo loro gli indirizzi politici all'interno della risoluzione. Ma questo non toglie la possibilità, a noi come Partito Democratico, di aggiungere delle riflessioni che accompagnano il nostro voto favorevole. lei va a rappresentare l'Italia, in un momento di difficoltà in cui la pandemia morde ancora, con la consapevolezza di aver fatto i compiti a casa. Ha ricordato giustamente, anche con una punta di soddisfazione (come è giusto che sia), la differenza dei dati di quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso. La campagna vaccinale con la terza dose ci pone più al riparo, incrociando le dita, rispetto agli altri Paesi

ci sono tante donne e tanti uomini che noi vogliamo ringraziare qui in quest'Aula, sanitari e non sanitari, persone dell'Esercito, volontari della Protezione civile che hanno permesso tutto questo. Da questo punto di vista, penso che stiamo dando un segnale importante con il progetto Covax, perché dà l'idea di come l'Europa sia anche l'Europa della solidarietà, che vuole mettere in sicurezza. Ed è giusto ricordare come l'Italia sia stata fra i primi a spingere per questo strumento e, allo stesso tempo, abbia lavorato per la centralizzazione degli acquisti e per costruire nuove regole a livello europeo. Adesso bisogna battere il ferro finché è caldo e costruire le condizioni per un'unione della salute; ne parliamo all'interno della conferenza sul futuro dell'Europa. Io penso che siano mature le condizioni per farlo a livello europeo, come a livello europeo ci sarà anche l'Eurosummit, l'occasione non solo per mettere in sicurezza l'unione bancaria, per completarla e dare stabilità e sicurezza al sistema finanziario, ma allo stesso tempo, all'interno di una dinamica dove siamo chiamati ad affrontare delle contraddizioni come quella di mettere più soldi, fare politiche espansive

Cambiare paradigma vale per il Patto di stabilità, che dovrà diventare patto di sostenibilità, ma vale anche sul tema della transizione energetica, dove affrontiamo tutte le contraddizioni della modernità, dei cambiamenti e della globalizzazione che ci entra in casa e ci cambia la vita. Questo vuol dire cambiare abitudini e fare un ragionamento franco, come quello che ha fatto lei, che certamente non è facile, sul tema delle rinnovabili e

a lavorare insieme, anche all'interno del Parlamento, per trovare risorse aggiuntive insieme al Governo sul caro bollette. Mi lasci dire che il Partito Democratico avrebbe visto di buon occhio la manovra anche sui redditi medio-alti, perché, nel momento in cui si chiede di più allo Stato, si chiede di più anche a chi può contribuire di più. *(Applausi)*. Da questo punto di vista non bastano certamente questi interventi contingenti, ma servono interventi strutturali a livello europeo, con gli stoccaggi strategici, ma anche un ragionamento sul prezzo

con il vicino russo bisogna trovare il modo di dialogare. Abbiamo apprezzato la sua telefonata e il confronto con il *Premier* russo; è una situazione in cui l'Europa si deve dimostrare molto ferma per evitare che venga messa in discussione l'integrità territoriale dell'Ucraina.

divisioni. Né ci possono essere divisioni dal punto di vista del fenomeno migratorio. Vorrei dire una cosa con grande chiarezza a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico su una vicenda che ci ha visto assistere a uno spettacolo indecoroso al confine fra la Bielorussia, i Paesi baltici e la Polonia. Sono giuste le sanzioni, è giusto essere sempre più duri nei confronti della Bielorussia e anche per questo il dialogo con la Russia è fondamentale. Penso però si debba anche spiegare ai *partner* europei che noi siamo diversi dai bielorussi, quindi anche ai polacchi bisogna dire in maniera molto chiara che ci sono delle regole in Europa, ci sono principi e valori che vanno rispettati *(Applausi)*. Noi i bambini che rischiano di morire sul confine li salviamo, perché in questo siamo differenti dagli altri

la natalità e la mortalità, rispetto a cui noi rischiamo di pagare un prezzo molto elevato, ormai dal 2013 non viene più colmato neanche dai flussi migratori, quindi da questo punto vista ci vuole

delle 5.000 persone che dovranno arricchire gli strumenti a disposizione dell'Unione europea. Quella forza, però, rischia di essere lettera morta se non investiamo su un'agenda politica condivisa, perché mentre noi esprimiamo solidarietà e siamo vicini ai baltici, ai polacchi, ragioniamo in termini di aiuti e di sostegni a quei Paesi, a volte non vediamo la stessa solidarietà e vicinanza quando chiediamo attenzione sulla rotta del Mediterraneo centrale, quando chiediamo più soldi sull'Africa subsahariana per la cooperazione: 6 miliardi per la rotta balcanica, neanche un miliardo per l'Africa. Bisogna spiegare a tutti i Paesi europei che noi discuteremo della riforma di Schengen, dei movimenti secondari, ma insieme vogliamo discutere della ridistribuzione obbligatoria, del *burden sharing* e del superamento del regolamento di Dublino, perché tutte queste cose si tengono insieme. Non c'è l'Europa *à la carte.* Si vince se si va avanti insieme. per non essere ipocriti e per non rispondere sempre con la frasetta per cui dobbiamo tutti lavorare insieme per passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata, dobbiamo anche cominciare a ragionare sul e a trattati vigenti rischiamo che questa partita non si possa giocare. L'enorme passerella non funziona, perché ci vuole unanimità; quanto alla stessa cooperazione rafforzata, i temi che riguardano la politica estera e difesa comune, come sa bene l'ex ministra Pinotti, Pinotti, hanno bisogno di una partenza condivisa da tutti i Paesi europei. Lei però, signor Presidente del Consiglio, sa benissimo quanto è stato difficile solo trovare una posizione comune quando si sparavano razzi dalla striscia di Gaza e da Gerusalemme, perché l'Ungheria ha alzato il ditino. Serve una modifica dei trattati, serve una convenzione: lo ha detto Scholz all'interno dell'accordo di programma che ha fatto partire il nuovo Governo. Dovremmo dirlo con forza anche dall'Italia: serve la modifica dei trattati e, parallelamente, la possibilità di agire anche fuori dai trattati. C'è chi vuole riprendere il sogno dei Padri fondatori: davanti alle grandi dei flussi migratori, dei cambiamenti climatici, della costruzione di un nuovo ordine internazionale, serve un'Europa unita e servono persone che abbandonino i propri egoismi e investano sull'Europa politica. Quindi facciamolo, o fuori dai trattati o con una convenzione. A chi sta Sta alla Francia, alla Germania e all'Italia. Oggi, con la credibilità del Presidente del Consiglio, tutto questo è possibile.

per prepararci insieme come Parlamento e come Paese agli appuntamenti della Conferenza sul futuro dell'Europa. Occorre anche capire insieme come si riscrive un patto in Europa, perché c'è la questione dei trattati, ma c'è un tema che oggi è fondamentale

l'Europa affrontasse nel suo insieme, anche con un meccanismo di solidarietà nuova, la crisi pandemica.

che non significa soltanto riscrivere il Patto di stabilità, che ormai si è consumato da solo e ha prodotto qualche danno, anche prima delle crisi. Oggi abbiamo la necessità di fare questo, come si vede dalla vicenda della della pandemia: se non applichiamo fino in fondo la solidarietà con i Paesi più poveri, se fino in fondo non superiamo anche la questione dei brevetti, non ci salviamo, perché adesso è Omicron,

che non abbiamo bisogno di chiacchiere a vanvera sul futuro del nucleare; abbiamo bisogno di fare, di intervenire, di investire e di essere tutti corresponsabili di una gestione democratica

dell'Europa la Polonia, per esempio, non faccia neanche intervenire le organizzazioni umanitarie per soccorrere e aiutare le persone. Questo non ci è piaciuto per niente.

Sappiamo bene, infatti, che il prolungamento dello stato di emergenza non è un fatto politico, ma nasce dalla necessità di non abbassare la guardia, di non perdere il vantaggio realizzato. Il Covid esiste ancora, in tutte le sue varianti. Finalmente lo stiamo gestendo, gestendo e non subendo, anche e soprattutto grazie alla struttura commissariale unita a tutto il personale medico, sanitario, scientifico, alla ricerca e alla campagna vaccinale efficace, oggi estesa anche ai minori, perché anche i minori si ammalano, anche i minori vanno a finire in ospedale e anche i minori sono fattore di contagio. Per questo, presidente Draghi, il Governo deve continuare e intensificare le corrette campagne informative per rassicurare le famiglie, per aiutare i timorosi a superare le paure. Ripeto, non possiamo perdere questo vantaggio proprio ora, vantaggio che sta salvando vite ogni giorno, che ci sta facendo tornare alla normalità. Lo stato di emergenza ha consentito di sostenere e aiutare ogni settore economico e sociale e adesso ha bisogno di un allunaggio morbido, perché si creino le condizioni per fare un passaggio delle consegne con una progressività che accompagni la ripresa con ordine e senza scossoni, anche perché all'emergenza sanitaria legata al Covid si sono aggiunte le emergenze economiche che ben conosciamo, legate ai temi degli approvvigionamenti energetici e delle materie prime. Come inoltre continuano a insistere i nostri coordinatori Tajani e Bernini, bisogna intervenire anche in maniera selettiva sulle cartelle esattoriali che incombono sugli italiani *(Applausi)*, aiutando chi in questo momento particolare non è in grado di assolvere ai propri debiti con il fisco, non perché inadempiente, ma perché non può. Consentitemi ancora, grazie a tutti la sua competenza e le capacità organizzative, ma, soprattutto, per le sue profonde doti umane. Ci congratuliamo per la sua meritata nomina a comandante del Comando operativo di vertice interforze, il COVI. Non dimentichiamo, come ha ben ricordato lei, presidente Draghi, che la buona gestione della pandemia e la campagna vaccinale massiva, come Forza Italia ha sempre sostenuto, in questa forma e con queste modalità, stanno consentendo all'Italia di recuperare e riprendere, portando il nostro Paese, da Paese vittima, a diventare Paese delle buone pratiche. Il modello Italia è preso ad esempio a livello europeo: vaccini e *green pass*; vaccini e *green pass* come strumento di libertà dalla malattia, per potersi muovere, incontrare e lavorare. Non ci stancheremo mai di ripeterlo e, come ha detto la presidente Casellati, se oggi l'Italia è davanti a tanti altri Paesi, non lo dobbiamo alla fortuna, ma alle scelte fatte in questi mesi, anche grazie al decisivo comportamento dei cittadini, che lei ha giustamente ringraziato. solo al tema più attuale, quello del Natale. In Italia abbiamo potuto realizzare i mercatini, consentire gli afflussi regolari nei negozi, nei ristoranti, negli alberghi, far salire al 100 per cento la capienza sugli autobus, mentre in molti altri Paesi europei tutto questo è ancora precluso e persistono le restrizioni. Penso a Paesi come Germania, Austria, Danimarca, Belgio, Regno Unito. Se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa, è a credere maggiormente in noi stessi e nella forza di reazione del nostro Paese. Noi non siamo secondi a nessuno. *(Applausi)*. Ci ha fatto piacere ascoltare i dati della nostra produzione e distribuzione dei vaccini oltre confine, che ci ricorda che dobbiamo allargare il nostro orizzonte, diventando protagonisti del sostegno vaccinale a livello mondiale, verso i Paesi più deboli, perché nessun Paese è un'isola e la pandemia deve sparire dalla faccia della terra, se vogliamo salvarci tutti. Questo vertice cui si accinge a partecipare, presidente Draghi, seppur di transizione, rappresenta un'occasione importante, che non va sprecata. A proposito di transizione, un tema importante che verrà affrontato è quello della transizione ecologica ed energetica, lo sappiamo. Si parlerà, del rincaro dei prezzi dell'energia, soprattutto per i Paesi dipendenti, come siamo ancora noi. L'aumento esponenziale e repentino delle bollette, mentre stiamo affrontando la rivoluzione verde, fatta di riconversioni e nuove formazioni per le imprese, si sta rivelando devastante e lo stesso per le Attenzione: l'Europa proiettata verso la neutralità climatica è la stessa che è ancorata al mondo delle energie fossili. Quindi, il sistema va affrontato con intelligenza e gradualità. Bene gli interventi a sostegno da lei illustrati per sollevare famiglie e piccole imprese da un peso insostenibile. Pensiamo al tema del gas e alle fonti rinnovabili. La ricerca, che è avanti in Italia, soprattutto per aprire al nuovo nucleare pulito, non è tempo sprecato. Bene la creazione di stoccaggi integrati di scorte di gas per far fronte ad aumenti imprevisti e la volontà di attuare rapidamente il terzo pacchetto del gas. L'attuale situazione del mercato elettrico non è perfetta, ma ci lavoreremo. L'Unione europea deve aumentare la flessibilità di rete, compresi lo stoccaggio, gli interconnettori, le reti intelligenti, la gestione della domanda. Poi c'è la questione della Russia e degli Stati Uniti. Insomma, ce ne sono tante. Ho sentito che metteremo in campo ogni iniziativa volta a favorire la distensione dei rapporti. Informazione e formazione per superare la sindrome da NIMBY e le paure legate alla non conoscenza e certezze sulle vie da da intraprendere, con uno Stato e un Governo amico. Forza Italia è un movimento europeista convinto, ma è anche un movimento liberale, che sta al fianco delle imprese, delle categorie produttive, del mondo del lavoro da loro generato. Vinceremo la sfida della transizione ecologica se riusciremo a governare i processi senza lasciare indietro nessuno: lavoratori e intere filiere di imprese. Indicare in maniera perentoria, come ha fatto il Comitato interministeriale per la transizione, nel 2035 il termine per la vendita delle auto con motore a combustione suona come un *ultimatum* e non come un'opportunità.

comunicazione della Commissione europea rispetto alla possibilità, per fortuna revocata, anche grazie all'intervento di Forza Italia e del PPE, di bloccare vendite e affitti per gli immobili che consumano. Continueremo a batterci. L'altra grande sfida è il passaggio definitivo da un sistema di economia lineare a uno di economia circolare, puntando a far diventare l'Italia da Paese povero di materie prime qual è sempre stato a Paese ricco di materie prime seconde. seconde. Vorrei chiudere sul tema dell'immigrazione. Il suo approccio umano, ma razionale è condivisibile. Dobbiamo stipulare un grande accordo con l'Africa, soprattutto del Nord, anche in tema di energie rinnovabili e ricordo il piano Marshall del presidente Berlusconi. Vorrei chiudere ribadendo

Forza Italia condivide il testo della risoluzione sottoscritta dai Capigruppo della maggioranza che la sostiene e, pertanto, nell'annunciare il nostro voto favorevole la invitiamo ad andare avanti sul cammino intrapreso perché il Paese ha bisogno di cura. Continui a curarlo come sta facendo.

presidente Draghi, abbiamo molto apprezzato la sua replica, più ancora che l'intervento iniziale, che sostanzialmente riprendeva quanto abbiamo ascoltato questa mattina nell'intervento alla Camera dei deputati.

Voteremo a favore della risoluzione che abbiamo steso insieme alla maggioranza che le dà degli indirizzi politici ben precisi attraverso i quali poter rappresentare in maniera compiuta l'interesse dell'Italia in sede europea. Nel suo intervento ha espresso che l'impegno del Governo non manca di coraggio e determinazione in un contesto difficile. Ne siamo pienamente consapevoli e questa è la stessa ragione per la quale ancora oggi siamo a dirle di andare avanti. Vada avanti finché ce ne sarà bisogno e dia tutte le risposte che il Paese si attende, senza trascurarne alcuna, a partire da quella che ci preoccupa molto relativa al carico molto relativa al carico fiscale che i nostri concittadini si trovano a dover sostenere tutto di un colpo perché rinvio dopo rinvio le scadenze sono arrivate, ma l'economia che dà significativi segni di ripartenza non mette ancora le nostre imprese e i nostri concittadini in grado di affrontare pienamente quelle scadenze. Occorre

la nostra voce su un problema serio all'interno del contesto europeo riguardo ai costi odierni dell'energia, ai costi che oggi le forniture relative al gas metano portano sia ai nostri concittadini che alle imprese. L'intervento del Governo è molto importante ed è apprezzabile nella sua dimensione volta a cercare di conservare il più possibile la capacità di acquisto dei nostri concittadini, ma c'è una dimensione che non può sfuggire

si trovano a dovere sostenere costi che hanno esorbitato oltre il 100 per cento rispetto all'inizio di quest'anno. Certamente 8 miliardi sono un intervento importantissimo. La sua affermazione precedente è pregna di realismo, ma proprio per questo occorre che ci sia una consequenziale azione del Governo,

con un approccio - e lo dico ai colleghi che compongono la maggioranza e anche l'opposizione - che non può e non deve essere ideologico, perché i numeri sono numeri, che siano scritti con la penna rossa, la penna nera o la penna blu. Ripeto che i numeri sono numeri e di tutto abbiamo bisogno, tranne che di un approccio ideologico su queste cose. Occorrono quindi pragmatismo e soluzioni che all'interno del contesto europeo non ci isolino, ma ci vedano, al contrario, protagonisti. Se per arrivare a questo protagonismo bisogna concludere anche nuovi accordi bilaterali, come quello che è stato fatto nei giorni scorsi con la Francia, bene, signor Presidente del Consiglio, vada in questa direzione nell'interesse dell'Italia. Ci siamo abituati troppo spesso a quel *refrain* per cui dobbiamo prendere decisioni nell'interesse dell'Europa. Abbiamo bisogno di tracciare la strada e se assieme a noi ci sono anche altri Paesi, bene: risvegli questa identità e porti all'interno del contesto europeo le nostre esigenze, non come marginali, ma come essenziali all'industria e al meccanismo economico del Vecchio continente.

Badi bene, non stiamo parlando di una cosa marginale, ma di qualcosa che da sempre, dal dopoguerra in avanti, ha trascinato lo sviluppo economico e la crescita nel Paese.

Anche questa volta, non vediamo una strategia europea, ma, al contrario, comunicati stampa che riprendono un po' per le orecchie l'Italia per le sue scelte, che possono essere più o meno condivisibili - lo vedremo *ex post* nei loro effetti - ma ma certamente tra la mancanza del fare e la scelta di fare, preferiamo chi sceglie di fare. Troppo spesso abbiamo visto l'Unione europea, come lei ha correttamente indicato, mancare nella sua decisione e non prendere decisioni efficaci sia in tema di politica estera, sia in tema di politica economica (una scelta economica fatta in ritardo è peggio di una scelta economica non fatta), ancora una volta in termini di contrasto alla pandemia. Signor Presidente, abbiamo fiducia che le azioni che il Governo sta mettendo in campo diano questi risultati siamo anche consapevoli che ci tocca fare qualche sforzo magari in termini di forma, apprezzando sempre quando il Governo viene prima in Parlamento e successivamente prende le decisioni, ma avendo ben chiaro che in situazioni eccezionali bisogna dare massima disponibilità. Anche in questa circostanza siamo qui a confermarlo. Tuttavia, signor Presidente, consentirà anche

Signor Presidente, ci consenta allora di mettere in evidenza che certamente non può essere una priorità del Governo quella del raddoppio della regolarizzazione dell'immigrazione clandestina; non può esserlo rispetto alle priorità che hanno gli italiani

corretta e leale né nei confronti di chi merita l'ospitalità, perché proviene da zone di guerra e deve essere protetto, né nei confronti dei nostri giovani, che vengono disincentivati a quello che nella Costituzione è riconosciuto come il fondamentale dei valori: il lavoro. Solamente nel lavoro ci sono l'uguaglianza, la fratellanza e la libertà. Su questi principi siamo certi, Presidente, che la sua azione all'interno del contesto europeo saprà essere pragmatica.

Anche in questo caso, il nostro aggancio al quadro atlantico non può essere messo in discussione, anche se in quest'Aula ci sono stati interventi che hanno strizzato l'occhio verso la Cina e quelle economie che altro non aspettano che una nostra flessione per potersi insidiare e poterci piegare. Non abbia dubbi a mantenerci ancorati al quadro atlantico, presidente Concludo in maniera molto semplice. Credo che, non a caso, alla fine del suo intervento abbia ricevuto un grande applauso. Può sembrare un applauso di circostanza; ebbene, Presidente, le rinnovo l'augurio di buon Natale che lei ha rivolto all'Assemblea, avendo ben chiaro che in questo suo augurio ci sono anche affermazioni di principio e d'identità che forse sono politicamente più rilevanti anche di tutte quelle che abbiamo fatto precedentemente.

Signor Presidente, presidente Draghi, colleghi, in questi due anni abbiamo fatto scelte importanti e consapevoli, basate sempre su evidenze scientifiche. Abbiamo fatto di tutto per porre fine a un dramma sanitario che è diventato anche economico e sociale.

come lei ricordava, Presidente), molti dei quali erano operatori sanitari. Abbiamo imparato a nostre spese cos'è la solitudine e abbiamo capito che la resilienza può fare miracoli. Adesso siamo all'ultimo miglio di questa, che è una maratona e non una corsa ai 100 metri, come abbiamo detto spesso, nella quale siamo sempre stati guidati dalla scienza, scienza, che è riuscita ad arrivare a un vaccino in tempi *record*, e noi, presidente Draghi, come ha detto lei, dobbiamo adottare ogni misura per evitare che il sacrificio sia stato vano. Allora, gli obiettivi devono essere quelli che abbiamo perseguito finora: salvare vite umane, mantenere bassa la pressione sugli ospedali e mitigare gli effetti economici di questa pandemia. Tutti vorremmo essere fuori da quest'incubo, ma le varianti che continuano a emergere richiedono cautela. Ci sono ancora troppi non vaccinati, ci sono troppe difficoltà per i Paesi poveri ad accedere ai vaccini. Il MoVimento 5 Stelle chiede da tempo di rivedere le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e l'accordo TRIPs e di liberalizzare i brevetti. Era il 1962, quando un medico polacco, che si chiamava Bruce Sabin, rinunciò al brevetto contro il vaccino per la poliomielite, quel vaccino che si somministrava con una zolletta di zucchero e che cambiò la storia dell'umanità. A chi gli chiedeva perché avesse rinunciato a quel compenso, Sabin rispondeva: i nazisti mi hanno ucciso due nipotine bellissime e allora ho deciso di fare questo regalo a tutti i bambini del mondo, perché non c'è uomo più potente di chi trasforma il proprio nemico in fratello. I vaccini, Presidente, sono lo strumento più potente che abbiamo per tenere basso il rischio sanitario. Anche il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz ha detto che non c'è ripresa economica, se non riduciamo il rischio sanitario. Lei, Presidente, dice spesso che non c'è ripresa economica, senza coesione sociale. Allora come rafforzare questa coesione sociale? A mio avviso, utilizzando tre strumenti. Il primo è la trasparenza la trasparenza nell'informazione che diamo ai cittadini per guadagnare sempre di più la loro fiducia. Il secondo è la partecipazione, perché i cittadini devono diventare attori protagonisti delle scelte di salute pubblica. Il terzo è la tutela dei beni comuni, ostacolando la logica del profitto a tutti i costi. Anche Papa Francesco, nella primavera del 2020, agli economisti riuniti a Cernobbio chiedeva di non sacrificare alla finanza la dignità della persona e di immaginare una nuova economia del prendersi cura della persona, un'economia della cura. con questi termi, la tutela dei beni comuni è al centro dell'agenda politica anche europea il MoVimento 5 Stelle ha avuto un ruolo determinante in questo processo di cambiamento. Il MoVimento 5 Stelle ha convinto l'Europa a passare da strumenti obsoleti, come il Meccanismo europeo di stabilità (MES), a nuovi strumenti di investimento, alimentati da debito comune e e condiviso *(Applausi)*, che sono il cuore del Next generation EU e del PNRR. È stato sospeso il patto di stabilità, si parla di superare il *fiscal compact*, è stato avviato l'acquisto centralizzato dei vaccini e si parla di salario minimo, di revisione del Trattato di Dublino, di difesa comune dei confini e di investimenti in fonti rinnovabili. Se avessimo avuto già da tempo questa visione di futuro, oggi non dovremmo correre ai ripari anche, ad esempio, per i rincari delle bollette. Infatti i dati dello UK Research Center e della Banca mondiale ci dicono che se investiamo un miliardo in fonti fossili, possiamo creare 9.000 nuovi posti di lavoro. Se lo stesso miliardo lo investiamo in fonti rinnovabili, creiamo 18.000 posti di lavoro, quindi il doppio. E allora questa è la strada: mettere al centro delle politiche, anche europee, la tutela dell'ambiente, della salute, del lavoro e dei beni comuni.

Grazie al MoVimento 5 stelle sono state introdotte misure come superbonus al 110 per cento, che stiamo ampliando e rafforzando nella legge di bilancio e che andrebbe esportato a livello europeo, perché sta guidando la crescita economica di questo Paese che quest'anno tocca il 6 per cento. *(Applausi)*. Ha creato 150.000 nuovi posti di lavoro, 70.000 nuovi cantieri, 30.000 nuove imprese. Il MoVimento 5 Stelle ha fatto partire le prime comunità energetiche, che sono luoghi di produzione, consumo e condivisione di energia. noi crediamo fermamente che il Governo italiano debba continuare in Europa ad essere promotore di questo percorso di cambiamento culturale che mette al centro la solidarietà, la responsabilità, la condivisione, la collaborazione e la tutela dei diritti umani. Il Governo dev'essere promotore di quella messa a sistema delle lezioni apprese dalla pandemia di cui lei parlava, parlava, che è stata un acceleratore di processi e ha avviato la transizione digitale (che non è solo utilizzare nuove tecnologie, ma migliorare i servizi), la transizione ecologica (che vuol dire ridurre il consumo per aumentare il benessere) e la transizione culturale (che mette al centro la persona). Se impareremo tutti a sacrificare un po' di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre ideologie e del nostro egoismo, potremo rafforzare in noi i nostri beni comuni, l'Europa

Signor Presidente, questo intervento le viene dall'opposizione di sinistra. Non è confortevole essere fuori dal *bias* cognitivo che ci governa e farsi fuori dalla narrativa generale, da questa pacata narrativa paternalistica. Personalmente, mi basterebbe credere al mezzo bicchiere pieno della collega Bonino, credere nell'Europa di cui si dice, improvvisamente diventata l'Europa dei popoli, e non vedere, ma bisogna resistere, difendersi dalle parole melliflue e guardare i fatti, vedere le politiche economiche *trickle-down*, che accrescono le differenze, le politiche repressive, divisive e falsamente persuasive, e vedere con occhio allenato il pacato negazionismo sui cambiamenti climatici e sull'ambiente. Non abbiamo fatto abbastanza - e questo è un fatto - per togliere i brevetti sui vaccini. Potremo farci quante dosi vaccinali vogliamo all'infinito, vaccinare i bambini e finanche i neonati, ma, fin quando i vaccini non saranno di libero accesso a tutto il mondo, non ne saremo mai fuori, visto che non possiamo mettere confini, alzare muri, sparare con gli idranti, affondare in mare o costruire barriere col filo spinato contro il virus. Contro il virus tutto questo non lo possiamo fare, come stiamo facendo invece con gli immigrati. *(Applausi)*. L'Europa sta facendo fare il lavoro sporco ad altri sui confini balcanici e sui confini confini con la Bielorussia, pacatamente condannando, ma accordandosi per il patto europeo per l'asilo, con l'intento di tenere tutti fuori dal nostro mondo ricco e sicuro. *(Applausi)*. Questa è la vostra resilienza? Quello che ci tocca fare è difendere il principio di asilo a qualunque costo, difendere il diritto internazionale e difendere i valori che ci hanno formato in qualunque condizione,

come in quello di Ponte Galeria, da dove ci giunge l'orrore della morte del giovane tunisino Wissem Ben Abdel Latif, non saremo mai l'Europa che ci raccontiamo di essere. *(Misto-IpI-PVU)*. Un Presidente del Consiglio senza mandato popolare, il Capo di un Governo profondamente tecnico ed elitario, sostenuto da una maggioranza che ha tradito il voto politico del 23 marzo 2018, va in Europa, cioè nel luogo meno rappresentativo degli interessi dei cittadini, a parlare per conto degli italiani, almeno così dice. Italexit per l'Italia questo mandato non glielo dà, perché non avete accettato, tra l'altro, la nostra proposta di risoluzione che chiedeva di bloccare le vaccinazioni ai bambini e di respingere ogni tentazione di obbligatorietà vaccinale. Per quel che ci riguarda, lei andrà al Consiglio europeo per difendere gli interessi di Big Pharma e del potere finanziario multinazionale che oggi punta le sue carte sullo *switch* energetico. Altro che normalità del Natale: voi state incattivendo vigliaccamente l'Italia con la propaganda dei buoni contro i cattivi. Più passa il tempo e più si fa palese la sudditanza dell'Unione europea e dei Governi verso Big Pharma. Un'inchiesta condotta dal «Financial Times» con Channel 4 dimostra, carte alla mano, l'asimmetria negoziale tra le istituzioni e la multinazionale americana che vende un vaccino concepito in Germania e pagato anche con i soldi del Governo tedesco. Un'inchiesta che dimostra la cattiveria di chi vi ha tenuto in scacco: avete permesso loro di fare quel che volevano, dalla segretezza dei contratti alla manleva totale, passando per la durezza delle contrattazioni sul prezzo dei sieri. Avevate detto che la cessione della sovranità nazionale serviva per costruire un'Europa forte nella globalizzazione. Invece, ancora una volta abbiamo la prova che le multinazionali e la finanza sono più forti del vostro baraccone europeo, lupo con i cittadini e pecorella al cospetto del nuovo ordine mondiale. i vaccini, Big Pharma dimostra il potere delle società quotate in borsa. Non a caso, parte dei profitti delle multinazionali del farmaco serve per attività di *lobby* nelle sedi europee. A proposito: la facciamo una Commissione di inchiesta seria sull'emergenza Covid, sui dati veri, su chi è pagato da Big Pharma, sullo scandalo delle mascherine e su tanto altro, o avete paura che vi scoprano? State ingrassando i bilanci di quell'1 per cento che divora il restante 99 per cento e lo fate con la solita propaganda dell'immunità, che non esiste. Il governatore dell'Italia Mario Draghi va in Europa con la cultura di Goldman Sachs e chi lo sostiene regge bordone a questa logica affarista e padronale, tanto che, a quanto pare, Draghi per la manovra non si farà neanche vedere in Aula. Complimenti governatore, buon Natale! Detto questo, a fare gli interessi delle multinazionali in Europa non ci andrà con il mandato di Italexit.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

e valorizzazione delle aree produttive ed industriali con l'esercizio di tutte le funzioni già attribuite ai singoli consorzi per lo sviluppo delle aree industriali tra le sue prerogative rientrava anche lo sviluppo dell'area industriale di Corigliano-Rossano (ex Corigliano calabro); tra il 2000 ed il 2004 nel territorio di Corigliano-Rossano decine di agricoltori sono stati espropriati dei loro agrumeti per pubblica utilità. Come risarcimento si offrì un prezzo irrisorio perfino al di sotto del prezzario agricolo. Per tale ragione nacque un contenzioso per la giusta determinazione del prezzo definito solo nel 2014 con sentenza della Corte di appello di Catanzaro; il CORAP, a fini dilatori, si oppose alla sentenza ma comunque la Corte di cassazione confermò la sentenza della Corte d'appello cristallizzando il diritto di credito degli espropriati e dunque la relativa indennità La Regione Calabria, invece di essere dalla parte dei proprietari, sta cercando di liquidare l'ente Corap, ma la liquidazione è stata giudicata illegittima dalla Corte costituzionale nel 2021. In questa disputa è intervenuto il Mise, che starebbe aiutando la Regione ad arrivare alla liquidazione; se questo dovesse avvenire, la Regione Calabria non pagherebbe gli espropri, in quanto la liquidazione seguirà le regole della *par condicio creditorum*. Il patrimonio della Corap però non è capiente e l'indennizzo dell'esproprio seguirà le regole del credito chirografario, con sicura beffa per gli agricoltori espropriati e mai indennizzati da oramai vent'anni. E' una situazione assurda e per questo motivo interrogherò il ministro Giorgetti, per capire se sia realmente a conoscenza della situazione e dei rischi che corrono i lavoratori della Corap, ma soprattutto anche gli ex proprietari mai indennizzati per i terreni espropriati da oramai vent'anni, che stanno aspettando il giusto risarcimento, con tanto di pronuncia da parte della giustizia amministrativa. La questione va risolta nel novero della legislazione vigente, perché, se gli ex proprietari non venissero pagati, oltre a rappresentare un'ingiustizia, questo episodio creerebbe un pericoloso precedente in materia di espropriazione. Ovvero, stando così le cose, lo Stato potrebbe espropriare e calpestare un diritto di proprietà, tutelato dalla stessa Costituzione, senza riconoscere una somma all'espropriato. *(Applausi)*.

cari colleghi, nell'agro sarnese-nocerino (e, precisamente, nella periferia di Scafati) accade che, a causa degli allagamenti che si ripetono da decenni, è diventato sempre più frequente che una comunità viva, anzi sopravviva, senza poter godere dei propri diritti, iniziando dalla libertà di movimento, fino al diritto a una giusta assistenza. Alcuni giorni fa, un'ottantenne, Maddalena Mandile, residente a Scafati, è morta, perché i soccorsi avrebbero subito rallentamenti a causa dell'acqua alta dovuta alle piogge (soccorsi che molto probabilmente le avrebbero potuto salvare la vita). Addirittura, a causa della strada allagata, anche il carro funebre ha avuto difficoltà a portare via la salma. Si tratta di una vicenda sulla quale tutti dobbiamo riflettere. La zona e questi allagamenti sono stati oggetto in passato di una mia interrogazione in Senato, oltre a ulteriori solleciti in Regione. In quella zona vanno immediatamente completati i lavori fognari e va effettuato un dragaggio dei canali; la Regione Campania, che è l'ente competente, deve intervenire al più presto, affinché le scene che ritraggono i residenti costretti a usare la barca per raggiungere la propria abitazione non si ripetano. Non si può morire così; non si può nemmeno vivere o, meglio, sopravvivere. Non si può, perché i residenti vanno tutelati. Non possiamo permettere che tali tragedie avvengano nel silenzio delle istituzioni. Cari colleghi e colleghe, dovete sapere che tutto l'agro sarnese-nocerino soffre di questi disagi. Le cause sono chiare e sono da ricercare nella mancata cura e messa in sicurezza del territorio. Peraltro, forse non tutti sapete che, a ogni pioggia un po' più intensa, le acque che provengono dal vesuviano scendono a valle, allagando puntualmente anche la stazione di Scafati e causando l'interruzione del trasporto pubblico su ferro in una tratta che va da città limitrofe, come Pompei, Poggiomarino, Sarno e Torre Annunziata, a Napoli. Concludo: lo Stato che rappresentiamo e la Regione Campania non possono più esitare. Bisogna intervenire al più presto e i lavori della rete fognaria devono proseguire spediti. Mi auguro che i rappresentanti regionali, di tutte le parti politiche, ascoltino questo mio appello. Ognuno di noi ha il dovere di essere vicino a chi vive questi disagi

La seduta è tolta